connotata da profili problematici e, soprattutto, da elementi di assoluta novità, che hanno imposto anche alla Giunta di condurre un'azione di approfondimento e di esame ancora più dettagliata e diffusa di quanto solitamente compiuto. Tanto è che, proprio in ragione di questi elementi, in questo procedimento si è registrata anche un'insolita evenienza, ossia un'interlocuzione tra la Presidenza della Giunta e la Presidenza del Senato in ordine ad una serie di aspetti Grazie, rispetto alla necessità di integrare la documentazione posta a disposizione della Giunta per l'esame complessivo. Questa insolita evenienza (cioè questa corrispondenza), tra l'altro tra l'altro occasionata proprio da una richiesta della Presidenza della Giunta alla Presidenza del Senato, ha permesso poi di delineare, nell'ambito delle conclusioni che sono state rassegnate, l'esatto schema procedimentale e soprattutto l'integrazione di quelle parti che sono risultate mancanti e rispetto alle quali, appunto, si è posta l'esigenza di un completamento e di un'integrazione. Dal punto di vista degli accadimenti e del fatto la vicenda non presenta aspetti particolarmente complessi, nel senso che tutto trae origine dalla registrazione di una trasmissione televisiva

Grazie, Pecorella, nella qualità di presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, e il dottor Edmondo Bruti Liberati, all'epoca presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Nel corso della trasmissione, l'onorevole Diliberto contestò la condotta del senatore Castelli, in modo particolare la circostanza che egli il giorno precedente aveva preso parte ad una manifestazione dei «giovani padani», ritenendo che nel corso della stessa fossero stati pronunciati *slogan* e assunti comportamenti non compatibili con la funzione ministeriale. In replica, il senatore Castelli, contestando la fondatezza del rilievo, muoveva rilievi più incisivi sulla condotta dell'onorevole Diliberto, in particolar modo sulla contiguità, per così dire, culturale e politica tra una rappresentanza parlamentare dell'estrema sinistra e taluni ambienti cosiddetti antagonisti che avevano dato luogo ad una serie di manifestazioni e di cortei durante i quali si erano registrati fatti di particolare violenza e, più in generale, tutto il clima che, in quegli anni, aveva connotato il dibattito politico su questi temi.

Correttamente l'autorità giudiziaria sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla Camera di appartenenza, in quel caso il Senato, per ottenere la pronuncia in ordine alla eventuale insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, sulle dichiarazioni che erano oggetto della contestazione e che avevano generato lo stesso contenzioso. In quella occasione, prima la Giunta, poi il Senato ebbero a deliberare nel senso di affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Castelli, quindi con la copertura della garanzia posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In quella circostanza già venne in evidenza un primo aspetto problematico della questione, vale a dire la protezione assicurata al parlamentare che contemporaneamente rivesta anche la carica di Ministro e rispetto al quale, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, intervenuta in materia di conflitto di attribuzioni, è possibile affermare l'insindacabilità quando sussista un nesso funzionale tra atti tipici del parlamentare e contenuto delle dichiarazioni che devono essere, secondo la giurisprudenza della Corte, sostanzialmente ripropositive nel contenuto di quanto affermato negli atti parlamentari. Rispetto a questa situazione, poiché il ministro-parlamentare non è nella condizione di porre in essere tutti gli atti tipici dell'attività parlamentare (si pensi, ad esempio, agli atti del sindacato ispettivo), sarebbe derivata - questo era l'avviso del Senato - una menomazione dello scudo, della protezione e quindi sostanzialmente anche una sorta di riduzione delle garanzie rispetto all'attività del parlamentare-ministro.

Rispetto a quel giudizio, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma rimise correttamente gli atti al collegio per i reati ministeriali (sempre presso il tribunale di Roma),

e quindi di rimettere la questione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per il proseguimento dell'azione penale.

ripose al Senato la questione relativa alla sindacabilità, questa volta *ex* articolo 68 della Costituzione, delle opinioni rese dal senatore Castelli. In quella circostanza, la Giunta delle elezioni ebbe modo di puntualizzare, in applicazione

parlamentare, non ci fosse necessità di una nuova delibera dell'Aula, potendosi ritenere che la precedente decisione del 30 giugno 2004

a prescindere da quale fosse stato successivamente il pronunciamento del Senato, che se il Senato avesse deliberato per la dichiarazione di insindacabilità andava comunque sollevato conflitto di attribuzioni.

la delibera della Giunta delle elezioni nella parte in cui richiamava la precedente delibera dell'Aula del 30 giugno 2004, in ordine alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Castelli. con una motivazione molto articolata, ma sostanzialmente incentrata sul profilo che la coincidenza in capo allo stesso soggetto della condizione di parlamentare e della qualità di Ministro, e quindi anche la limitazione delle funzioni parlamentari (un esempio tipico è la non proponibilità degli atti di sindacato ispettivo), non non costituisse ragione per ritenere estensibile al di là del nesso di stretto collegamento funzionale la tutela *ex* articolo 68, nonostante, appunto, al Ministro sia, per previsioni del Regolamento della Camera di appartenenza, precluso il ricorso a tutta una serie di atti tipici. Quindi, questa riduzione non rappresenta, ad avviso della Corte, per sovvertire o modificare quel consolidato orientamento giurisprudenziale dalla stessa formato attraverso una serie ripetuta di pronunce in ordine alla rigorosa applicabilità del criterio del nesso funzionale. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale il senatore Castelli pone una serie di questioni, in particolar modo in ordine alla ministerialità del reato e, soprattutto, sulla ricorrenza dell'esimente *ex* articolo 9, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, questioni che sono state diffusamente illustrate anche nella relazione della Giunta e che si incentrano sostanzialmente sulla latitudine del concetto di reato ministeriale accolto dopo la novella del 1989 nell'articolo 96 della Costituzione, sulla erroneità, per così dire, della pronuncia dell'ordinanza del tribunale dei ministri che motiva il diniego del carattere di ministerialità argomentando dall'articolo 68 sull'insindacabilità e dunque su materia che non è di competenza del tribunale dei ministri e che non ha alcuna influenza in ordine alla ricorrenza della ministerialità, e soprattutto rispetto alla funzione delle dichiarazioni che sono state rese dal senatore Castelli nell'esigenza di tutelare l'azione del Governo e le scelte legislative fatte dallo stesso in campi particolarmente sensibili, quali la lotta al terrorismo e la riforma dell'ordinamento giudiziario, che impegnano politicamente il Governo, che hanno rilevanza costituzionale. In questo senso la Giunta, a maggioranza, ha rassegnato le sue conclusioni di ritenere il carattere ministeriale del reato e la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, di avere agito il Ministro del tempo per la protezione e la tutela di un preminente interesse nazionale nella funzione di governo.

Grazie,

il quale ha invitato tutti gli organi istituzionali, tutte le forze politiche, ad evitare scontri, conflitti di qualsiasi genere e ad abbassare i toni. toni. In questa materia è già intervenuta la Corte costituzionale due anni fa, nel luglio del 2007, in relazione ad un conflitto che era stato sollevato, come ha ben ricordato il relatore, tra il Senato della Repubblica e il tribunale di Roma, già due anni fa la Corte costituzionale aveva dato torto al Senato e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, annullando una deliberazione della Giunta e restituendo gli atti al Senato. Si trattava dello stesso caso per quanto riguarda la persona del senatore Roberto Castelli e si tratta ora di un problema diverso che viene proposto all'esame di questa Assemblea. Il relatore ha illustrato i fatti che stanno alla base di tale questione e quindi non mi dilungo sulla vicenda da un punto di vista storico. Segnalo, peraltro, che è già stato richiesto l'intervento della Corte costituzionale in una situazione giuridica analoga, che è quella che riguarda l'allora ministro dell'ambiente Matteoli, e a questo proposito la Corte costituzionale, in data 9 luglio di quest'anno, ha annunciato via stampa l'accoglimento del conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale dei ministri di Firenze

la motivazione di decisione del 9 luglio dovrebbe essere depositata a giorni. Ovviamente, questa nostra richiesta sospensiva non ha alcun intento dilatorio, ma vuole soltanto essere utile ai lavori del Senato, anche perché sulla base della motivazione che verrà depositata, e quindi sulla base delle indicazioni giuridiche della Corte costituzionale, è possibile che il Partito Democratico decida di votare in un senso oppure nell'altro, prendendo atto dei princìpi giuridici che saranno segnalati e scritti dalla Corte costituzionale. Pertanto, proprio nell'ottica segnalata dal Presidente della Repubblica, per evitare conflitti e contrasti istituzionali di altissimo livello e per evitare che ancora una volta la Corte costituzionale intervenga e dia torto al Senato in una materia così delicata, chiediamo che l'Assemblea

davvero credo sia venuto il momento di porre la parola fine su questo caso e di decidere questa mattina in merito alla proposta del senatore Sarro, contenuta nell'ambito di una relazione sicuramente articolata e densa di argomenti tecnico-giuridici a favore dell'accoglimento della proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Castelli. La proposta di questione sospensiva illustrata poc'anzi dal senatore Casson ovviamente ha un intento meramente dilatorio: il caso Matteoli è stato sottoposto al giudizio della Corte, la quale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni, però non ne conosciamo ancora le motivazioni;

Costituzione. In realtà, nell'ambito della Giunta - e la relazione del collega Sarro è molto precisa anche su questo punto (in particolare, il senatore Sarro fa riferimento specifico anche alla contemporanea presenza di un giudizio dinanzi alla Corte sul caso Matteoli) abbiamo già dato una lettura costituzionalmente orientata di queste disposizioni e abbiamo quindi indicato una linea necessitata di valutazione di questo caso, che ci porta a ritenere assolutamente infondata questa richiesta di sospensiva. Dunque, esprimiamo un giudizio negativo nei confronti della richiesta di rinvio della trattazione di questo argomento. Concludo dicendo che il principio di leale collaborazione, che prima citava il collega Sarro, tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria ordinaria,

e non certo per colpa del Parlamento, del Senato della Repubblica. Il procedimento penale oggi pendente dinanzi al tribunale di Roma è stato caratterizzato da anomalie, da ambiguità sin dagli inizi. Dunque, siamo oggi chiamati a porre un freno a queste anomalie, a ricondurre questo procedimento nel binario corretto della democrazia.

La medesima vicenda, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico e costituzionale,

potrebbe far intendere che il tipo di decisione sia nel senso delle conclusioni cui è pervenuta la Giunta nella sua valutazione, costituzionalmente orientata. Il problema è che leggere le ragioni dell'accoglimento del profilo di costituzionalità implica diversi aspetti: può significare che, qualora si proceda all'archiviazione in caso di reato non di competenza del tribunale dei ministri,

può, invece, dirsi che la comunicazione alla Camera di appartenenza, in linea con le altre comunicazioni che devono essere date in tutte le ipotesi di archiviazione, debba farsi in quanto abiliti in questo modo la Camera di appartenenza a decidere essa della ministerialità o meno noi non sappiamo quale delle due decisioni la Corte costituzionale condivide. Se la Corte costituzionale condividesse esclusivamente l'obbligo, contenuto nella legge del 1989, di comunicare alla Camera di appartenenza la conclusione del giudizio

se invece la decisione fosse nel senso che la comunicazione può ovvero deve introdurre la procedura che oggi qua stiamo trattando, allora avrebbe ragione la Giunta nella sua proposta nella sua proposta odierna. In queste condizioni, trattandosi di una decisione il cui contenuto conosceremo di qui a pochi giorni, perché commettere un errore? Aspettiamo alcuni giorni, sapremo come la Corte costituzionale ha interpretato le norme e ci adegueremo ad esse, senza dover per forza divinare ciò che la Corte ha scritto nel provvedimento, perché obiettivamente non siamo in grado di saperlo. Ritengo quindi fondatissima la richiesta di sospensiva proposta, alla quale il nostro Gruppo voterà favorevolmente.

vi sta presentando rappresenta per molti di noi, che hanno lavorato per parecchio tempo a questo caso, un atto che non esitiamo a definire abnorme,

molto severo. Ci troviamo di fronte ad una questione in se stessa abbastanza poco significante, una di quelle che normalmente vengono trattate dal Senato della Repubblica nell'ambito del giudizio di insindacabilità parlamentare delle opinioni espresse dai senatori.

I due se le sono date di santa ragione, politicamente, come tante volte accade in un dibattito televisivo, al termine del quale il ministro Castelli,

e che quindi il senatore Castelli doveva essere normalmente sottoposto al giudizio ordinario, come tutti i cittadini italiani. Peraltro, questo succede molte volte,

il funzionamento del Parlamento, quando è chiamato ad essere in qualche modo giudice di se stesso. È tutto ciò che è avvenuto dopo che definisce in termini di anormalità quanto si sta proponendo di votare.

è diventato improvvisamente un giudizio richiesto su una pretesa condotta del senatore Castelli come ministro della giustizia. Sono due casi diversi. Questo secondo è disciplinato dall'articolo 96 della Costituzione, in cui si dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono giudicati dai tribunali ordinari, previa autorizzazione della

a valutare se la *notitia criminis*, cioè la condotta attribuita al Ministro, è configurabile come reato è una sezione speciale del tribunale, il cosiddetto tribunale dei ministri, che funge sia da pubblico ministero che da giudice per le indagini preliminari.

di quella che viene definita giustizia politica, per cui, a un certo punto, non è più un giudice ordinario ma l'Assemblea parlamentare a giudicare il Presidente del Consiglio o i Ministri abbiano commesso quei fatti nel perseguimento di un preminente interesse pubblico e nell'esercizio della funzione di governo. A quel punto, se quest'Aula se quest'Aula decidesse che questo preminente interesse pubblico esiste ed è stato perseguito nell'esercizio di un'azione di governo e non nell'esercizio di un'azione da privato cittadino, da parlamentare,

Il tribunale dei ministri ha dichiarato al Senato che intende giudicare il ministro Castelli perché ha commesso un reato ministeriale? No, non è successo questo. È successo che il tribunale dei ministri ha stabilito che partecipare ad una trasmissione televisiva in cui ci si azzuffa tra uomini politici,

un corretto adempimento dei doveri da parte del Collegio per i reati ministeriali, e questo era oggetto di una valutazione della Corte costituzionale. Non abbiamo voluto né vogliamo attendere la sentenza che ci spieghi come procedere in questo caso di declinata competenza del tribunale dei ministri. punto rimane l'altra strada, cioè quella di giudicare secondo quanto prevede la Costituzione e la legge costituzionale. L'abbiamo fatto? Lo dico chiaramente: non l'abbiamo fatto.

per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Mi vedo costretto a ricordare che noi non abbiamo visto nulla dell'indagine condotta dal tribunale dei ministri, che nessuna

dalla Costituzione alla nostra funzione di parlamentari e anche in quella che garantisce il lavoro dei Ministri e del Presidente del Consiglio, ma declassarla Presidente del Consiglio, ma declassarla ad impunità per questioni che possono essere, magari con maggior successo, difese secondo

*(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'abolizione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari è venuto meno un fondamentale bilanciamento nell'equilibrio tra i poteri, ma si è aperta anche - e purtroppo - una surrettizia rincorsa a dilatare altri istituti giuridici per conseguire come risultato la tutela del ceto politico quantomeno simile. Non solo sono contrario a questo modo di procedere, che non riconosce la dispersione venutasi a creare sotto l'impulso della piazza ma surrettiziamente cerca di riguadagnare terreno, ma sono altresì convinto che esso dia luogo a vistose disparità di trattamento, gravi anomalie procedurali e possibili conflitti con altri poteri dello Stato. Infatti, in luogo della leale collaborazione richiesta più volte dalla Carta costituzionale, viviamo quotidianamente una fuga dal processo nella quale alcuni studi legali si sono specializzati operando nelle pieghe del sistema giuridico. Il presidente Follini ci ha già ricordato qualche mese fa come ciò avvenga con lo scudo di cartone rappresentato dalla dilatazione della insindacabilità parlamentare. Mai avremmo immaginato però che ciò potesse raggiungere le forme atipiche di una procedura vistosamente abnorme che attinge dalla presunta natura ministeriale di un reato commesso da un parlamentare. La Corte di cassazione è chiarissima nell'evidenziare che non basta il requisito soggettivo di appartenenza al Governo, ma occorre anche una connessione oggettiva con le funzioni svolte. Qui, invece, nulla può considerarsi riferibile (almeno per gli atti che abbiamo avuto la ventura di leggere) alla competenza funzionale del Ministro della giustizia del tempo. Eppure, è proprio questo che da oltre otto mesi sostiene la maggioranza. Se vi pare che la libertà di critica del parlamentare sia compressa, cari colleghi, ripensiamo insieme all'articolo 68 della Costituzione! Non cerchiamo scorciatoie o forzature: infatti, non è una soluzione quella di travestire l'espressione della critica con una presunta natura ministeriale e, meno che mai, con una esimente immaginata per gravissimi motivi di ordine generale. Invece di riequilibrare la bilancia tra i poteri (Parlamento, Governo, magistratura), qui si vuole tutelare soltanto una parte e, nell'ambito della parte (i Ministri), solo alcuni (quelli della maggioranza in essere). L'effetto distorsivo di tutto ciò è evidente: se il Parlamento può dichiarare la ministerialità del reato in dissenso dal tribunale dei ministri, è possibile anche l'opposto, che il Parlamento sottragga lo scudo della procedura ministeriale ad un soggetto che in astratto ricadrebbe nell'articolo 96 della Costituzione. Un Ministro di altra legislatura ed altra maggioranza potrebbe, in base a tale decisione, vedersi privato della possibilità di andare esente da pena, in ragione di una stretta disciplina di maggioranza diversa da quella che lo espresse come Ministro. Quel che è peggio è che la procedura escogitata, in questo caso, ha offerto ulteriori corollari aberranti: lo stesso diritto di difesa - imposto dalla legge costituzionale e dall'articolo 135-*bis* del Regolamento per la procedura di valutazione dell'esimente - non è stato applicato per la valutazione della ministerialità. Debbo lamentare una grave lacuna procedurale, onorevoli colleghi, che nessun avallo della Presidenza del Senato può arrivare a sanare: il senatore Castelli non è stato ascoltato, a dispetto delle previsioni di legge e di Regolamento. Questo precedente diventerà lesivo se e quando, in futuro, la ministerialità sarà esclusa a dispetto della pronuncia giudiziaria e della volontà dell'interessato. Comprendo lo scrupolo con cui la Presidenza della Giunta ha svolto, egregiamente, il suo ruolo istituzionale, dando esecuzione alle istruzioni - per la verità, un po' troppo pedisseque - pervenute dalla Presidenza del Senato. Debbo però lamentare che tali istruzioni hanno avuto scarso riguardo per i princìpi processuali e costituzionali fondamentali, come quello del contraddittorio, cui ho già fatto riferimento, e quello della completezza della cognizione, in totale assenza di atti processuali. colleghi, l'inseguimento delle vicende processuali da parte della maggioranza della Giunta ha impresso una forzatura non rimarginabile ai lavori; ad ogni udienza del dibattimento penale, dinanzi al tribunale di Roma, la maggioranza ha fatto precedere o seguire un'iniziativa di impulso in Giunta. Su tutto ciò voglio essere chiaro, da testimone presente ai lavori della Giunta. Voglio dare atto della correttezza dell'operato del presidente Follini e dei suoi Uffici; non riconoscerlo oggi significa aprire una breccia nella quale la certezza del diritto, la funzione di garanzia e la salvaguardia delle procedure sono destinate a soccombere. È tutto sommato indifferente che le forzature della maggioranza siano finalizzate a precostituire un precedente a favore di futuri casi o invece servano solo a facilitare la difesa tecnica di avvocati privi di ulteriori argomenti e, se mi è consentito, anche di ulteriori scrupoli. La cosa rimarchevole è, invece, che ne discende l'alterazione della tranquillità decisionale dei magistrati che conoscono del caso del senatore Castelli in sede giudicante, lasciando intendere che sia imminente una "valutazione insindacabile" del Senato sull'oggetto del loro giudizio. loro giudizio. Porre la reputazione di un rivale politico al di fuori dell'interesse pubblico è innovazione assai grave; ancora più grave è cambiare i procedimenti previsti dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari solo per un singolo caso, consolidando pericolosissimi precedenti. Se l'interesse pubblico è quello di una parte, rischiamo di consacrare a favore di chi, provvisoriamente, governa - una predominanza che esclude, per il contraddittore, la possibilità di chiedere tutela giurisdizionale. L'esercizio della funzione di governo avviene a nome di tutta la collettività nazionale, e non solo di una parte. Anche il riconoscimento dell'esimente dovrebbe essere svincolato da una succube concezione di stretta maggioranza, a fronte della quale le procedure sono viste come un incomodo impaccio. Ma c'è ancora oggi chi, per vezzeggiare il suo elettorato antipolitico, racconta solo una parte della verità: l'articolo 68 della Costituzione resta quello imposto dalla nefasta stagione di Tangentopoli, e poi surrettiziamente si dilatano gli istituti giuridici esistenti, per addivenire ad una copertura impropria di comportamenti estranei alla loro stessa *ratio*. Tutto ciò mi pare un segnale di serio degrado della cultura politica del nostro Paese. Tali gravissime ricadute della proposta approvata dalla maggioranza della Giunta mi inducono ad annunciare che non prenderemo parte alla sua votazione. Si tratta, infatti, di una procedura che, a prescindere dalla valutazione di merito sulla posizione del collega Castelli, è totalmente al di fuori della Costituzione, delle leggi che regolano la responsabilità ministeriale e dei nostri Regolamenti; una procedura surreale che con il nostro voto non possiamo contribuire a stabilizzare come precedente per quest'Aula.

e, quindi, l'impossibilità per l'allora ministro Castelli di fare ricorso a tale qualificazione giuridica. Il senatore Castelli, allora ministro, nella ricordata lettera del 30 ottobre 2008 afferma che durante la trasmissione televisiva in cui fece le dichiarazioni oggetto del giudizio subì, da parte del deputato Diliberto, attacchi aventi ad oggetto la sua funzione di Ministro della giustizia e la riforma da lui proposta in materia, nonché la funzione di Ministro della Repubblica, con l'accusa di aver compiuto, durante una manifestazione, atti non compatibili con la stessa. Afferma il senatore che solo in risposta a questa accusa, inerente le sue funzioni ministeriali, egli pronunciò le frasi in questione, che erano comunque da ritenere strettamente connesse con le attività di Ministro. Il senatore Castelli conclude la sua memoria dicendo: «Appare quindi evidente che il mio intervento nei confronti dell'onorevole Diliberto era correlato allo svolgimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo nel difendere, anche con toni forti, una riforma della giustizia che il Governo aveva presentato e fatto approvare e che riteneva di assoluta rilevanza per la vita del Paese». Il senatore Castelli faceva questo riferimento perché, in effetti, solo due sono i motivi per cui il Senato può negare un'autorizzazione a procedere. Faccio riferimento alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, laddove si dice

rilevante, ovvero nel perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Non sembra proprio che queste indicazioni abbiano a che con fare il caso di specie. Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata della previsione dell'articolo 96 della Costituzione limita l'ambito di applicazione della speciale procedura da essa prevista ai reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni. A questo proposito, fin dal 1994 le sezioni unite della Corte di cassazione ebbero modo di rilevare, con riferimento alla fattispecie, che la Costituzione, evitando una specifica previsione di singole fattispecie di reato, ha preferito fare riferimento a tutte le ipotesi di reato ravvisabili nell'ambito dell'ordinamento positivo dello Stato, sicché gli elementi qualificanti della previsione sono affidati alla concorrente presenza di due circostanze: la particolare qualificazione soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal Ministro.

l'avvertita esigenza di utilizzare criteri riduttivi per limitare l'eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria, è sufficiente fare ricorso ai risultati interpretativi a cui la Corte di cassazione (così sempre parlano le sezioni unite) è pervenuta in relazione a tutte quelle ipotesi di reato nelle quali la condotta incriminata richiede un rapporto di condizione strumentale con l'esercizio di determinate funzioni. Fa riferimento, ovviamente, ad articoli specifici e reati contro la pubblica amministrazione. Così continua la Corte: «Nell'ambito di tutte queste numerose fattispecie si è sempre affermato che, con l'espressione "esercizio delle funzioni", il legislatore ha inteso fare riferimento alla competenza funzionale dell'autore del fatto, sicché il rapporto strumentale connessione sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto». Da ciò discende ovviamente che, così come il nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni non può essere equiparato a un rapporto di oggettiva connessione, altrettanto arbitrario sarebbe arricchire quel rapporto di ulteriori elementi qualificanti, come l'abuso dei poteri o delle funzioni o la violazione dei doveri di ufficio non richiesti dalla legge, né suggeriti da una corretta interpretazione. Quindi, soltanto il rapporto oggettivo e strumentale con l'esercizio delle funzioni è il criterio utilizzabile per la delimitazione della categoria dei reati ministeriali. È evidente che il caso di specie è totalmente diverso. Si tratta della semplice partecipazione dell'allora ministro Castelli a una trasmissione televisiva. descritta dell'onorevole Castelli ... è ... totalmente estranea all'esercizio delle sue funzioni di Ministro della giustizia, in quanto la trasmissione televisiva in cui sono state rese le dichiarazioni di cui aveva ad oggetto il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario ed era ormai al termine e le dichiarazioni non hanno alcun nesso funzionale con atti tipici parlamentari, con la qualifica istituzionale rivestita dall'onorevole Castelli,

intervenuto su questa vicenda. Non è dato, infatti, invocare in questa situazione nemmeno l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di eventuale giudizio penale rese nel corso della predetta trasmissione televisiva, in quanto difetta addirittura - come come diceva il tribunale - quella corrispondenza sostanziale di significati tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle rese in una sede esterna, che sola può giustificare la garanzia dell'insindacabilità. Tanto meno - si dice e sosteniamo - è prospettabile un richiamo in questo caso ai privilegi garantiti a un Ministro della Repubblica dalla nostra Costituzione. Ripeto, si tratta della semplice partecipazione ad un confronto televisivo. Allora, non basta avere i sottotitoli della trasmissione che che indicano che l'oratore è un Ministro per poter invocare la speciale procedura prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989. Se si fa politica in una trasmissione televisiva e se si accetta il contraddittorio in quella sede, non si può e non si deve ricercare un piano privilegiato di tutela, magari per poter dire qualcosa in più rispetto ai propri interlocutori. della giustizia Castelli voleva accettare il dibattito tra pari, forte solo delle sue idee, non deve ora ricercare uno scudo con il quale evitare di difendersi dall'accusa di diffamazione. Questo scudo non gli è riconosciuto, in quanto la giurisprudenza prevede che sia ministeriale il reato commesso in rapporto oggettivo e strumentale con l'esercizio delle funzioni di componente del Governo. Questo rapporto non c'era nella trasmissione televisiva e per questo motivo è giusto che il senatore Castelli oggi si difenda dall'accusa rivoltagli dall'onorevole Diliberto in tribunale, senza che il Senato entri in alcun modo nella controversia. Se il Senato, invece, accoglierà la richiesta dell'allora ministro Castelli, significherà scegliere di estendere il piano dei privilegi aggirando norme costituzionali, creando un grave *vulnus* alla nostra Carta costituzionale allontanando, di conseguenza, sempre di più i cittadini dalla classe politica e di governo, che sarà vista sempre di più come casta intoccabile, che in caso di pericolo si autoassolve e che nega soltanto per sé stessa il rispetto dovuto alle leggi,

in base al quale il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari gli atti gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

il Senato per non avere, nel 2005, affrontato il problema nell'ottica dell'articolo 96 e si chiedeva, nel 2008, ciò che il Senato aveva ritenuto di non fare nel 2005. nel 2005. Il caso è proprio al di fuori del Regolamento. Noi non abbiamo ricevuto dall'autorità giudiziaria alcun atto. Come si innesta la procedura che stiamo applicando? L'autorità giudiziaria non ha chiesto di poter processare il senatore Castelli per un reato ministeriale, per cui si applicherebbe l'articolo 135-*bis*, in quanto non ritiene che si tratti di un reato ministeriale. Allora, di cosa dobbiamo occuparci? Del fatto che il senatore Castelli chieda che il reato che si ipotizza a suo carico sia di natura ministeriale? Lo chiede lui?

nella lettera della Presidenza del Senato dell'11 gennaio 2006, protocollo n. 7610,

«sono peraltro dell'avviso che tutto il sistema delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'autorizzazione a procedere per i cosiddetti reati ministeriali presuppone l'iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente e non può essere attivato su richiesta anche se, come in questo caso, perfettamente giustificata - dell'interessato». Questo è il precedente che abbiamo. Tale procedura non può essere attivata su richiesta dell'interessato, ma presuppone,

strano. È stata attivata una procedura iniziata con gli atti della lettera del senatore Castelli alla Giunta

Può oggi il Senato pronunziarsi su qualcosa che escluse di fare in passato? Si obietta che il Senato non sapeva ufficialmente che esistesse una pronunzia del tribunale dei ministri che aveva ritenuto non ministeriale il reato. Non è vero: il Senato lo sapeva benissimo, tanto è vero che si è costituito innanzi alla Corte costituzionale nel giudizio promosso dall'autorità giudiziaria, che lamentava il giudizio del Senato in base al quale aveva ritenuto insindacabili, e quindi coperte dall'articolo 68 della Costituzione, le dichiarazioni e le affermazioni del senatore Castelli. Quel giudizio fu introdotto dalla magistratura, che poi ebbe ragione, perché la Corte costituzionale dichiarò che il Senato aveva sbagliato a ritenere insindacabili quelle dichiarazioni.

in considerazione della carica ricoperta dal senatore Castelli nel Governo, aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto la restituzione degli atti, ritenendo che si trattasse di reati comuni».

il Gup del tribunale di Roma ha notificato il ricorso e l'ordinanza al Senato della Repubblica in data 21 febbraio 2006

chiedendo che (...) il ricorso sia dichiarato inammissibile e, nel merito, che la Corte statuisca - accertato che i fatti per cui è in corso procedimento penale di fronte al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma

di incompetenza del tribunale dei ministri, tant'è che nell'atto di costituzione innanzi alla Corte costituzionale non sollevava alcun profilo:

costituzionale n. 1 del 1989, ossia che «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo». Qual è il fatto

di avere, dinanzi al Palazzo del Senato, il 17 marzo 2004, saltellato al grido «chi non salta, italiano è». Il ministro Castelli risponde: «piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltare». Questa è la vicenda. Oggi il senatore Castelli dice che intanto ha risposto in questa maniera aggressiva all'onorevole Diliberto, che lo aveva accusato

un'attività tipica ministeriale e se rientri nelle prerogative del Ministro, sicché per difendere tale prerogativa gli sia consentito di aggredire chi lo accusa di averlo fatto. Poniamo il caso paradossale che colui che salti, nel ricadere in terra, si imbatta nella caviglia di un ignaro cittadino procurandogli una lesione, che si instauri un procedimento per lesioni colpose: dobbiamo ritenere questo fatto un reato ministeriale? *(Applausi

oppure, secondo quanto viene proposto, «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo»? Siamo al ridicolo! Si chiede che il saltellare gridando «chi non salta italiano è», ossia il contrario dell'essere Ministro della Repubblica italiana, sia considerato esercizio di una funzione ministeriale esercitata «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico». Mi rifiuto di prendere in considerazione una decisione del Senato che voglia assegnare a tale vicenda la sacralità del ruolo che i reati ministeriali assumono e che li porta ad essere così rigorosamente valutati, disciplinati e decisi! Ritorniamo con i piedi per terra.

e, in particolare, che chiamano in causa sotto questo aspetto il Governo, la maggioranza e il Parlamento. Soprattutto dal Parlamento, probabilmente, il popolo italiano si aspetterebbe qualcosa di più, e in questo caso non la difesa di una casta. Credo che i colleghi che mi hanno preceduto abbiano posto in rilievo molti argomenti che richiederebbero un'attenta riflessione e soprattutto una risposta da parte del Senato, oggi, che sia assolutamente diversa da quella che finora è stata data. E non soltanto perché la Giunta ci pone un problema e ci chiama davvero a pronunziarci come Assemblea sulla declaratoria del carattere ministeriale del reato, ma perché mi sorprende che il Senato si sia rifiutato questa mattina di sospendere la decisione in attesa

Segue un procedimento penale, rispetto al quale vi è una pronunzia di incompetenza del tribunale dei ministri con conseguente trasmissione degli atti

A seguito di quanto avvenuto viene investita nuovamente la Giunta, la quale dichiara che non c'è luogo a procedere, e viene sollevato un conflitto di attribuzioni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 10 luglio 2007, si pronunzia riattribuendo al giudice ordinario i suoi poteri,

gli ammonimenti del Presidente della Repubblica, che in questo periodo cerca disperatamente di difendere la Costituzione e di richiamare i poteri dello Stato ad una lealtà nei loro rapporti. Credo che mai come in questo caso ci dovrebbe essere una lealtà nei rapporti tra i diversi poteri dello Stato. seguito dalla Giunta è del tutto anomala. Infatti, come giustamente è stato ricordato dai colleghi, non è il tribunale ministeriale che dichiara di voler procedere nei confronti del senatore Castelli (anzi lo esclude), ma è il senatore Castelli che, attraverso una lettera che in maniera del tutto irrituale viene inviata al Presidente del Senato e da questi trasmessa alla Giunta delle elezioni chiede di essere considerato responsabile di un reato ministeriale. Credo che più abnorme di così non potrebbe essere l'*iter* che viene sottoposto alla nostra attenzione. chiede quindi che quel suo comportamento, tenuto in una trasmissione televisiva, sia considerato un fatto di «preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo», di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tutto questo in totale violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto,

prevista per i reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni deve avere una interpretazione assolutamente restrittiva. Non è possibile attribuire all'occasionalità del fatto la valenza di reato ministeriale. Alterare questa qualificazione giuridica, come è successo nel caso che stiamo esaminando, finirebbe per rappresentare, tra l'altro, un pessimo uso delle attribuzioni parlamentari del Senato, perché sostenere che vi sia un fatto di preminente interesse di preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo in un diverbio tra il senatore Castelli e un avversario politico è davvero qualcosa di inqualificabile. Tutto questo quando la giurisprudenza ha messo in luce - e mi sembra molto sensatamente - che «il carattere politico del reato, il movente che ha determinato il soggetto a delinquere, nonché il rapporto che può sussistere tra il reato commesso e l'interesse pubblico della funzione esercitata, proprio in conseguenza di quanto disposto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono criteri idonei a giustificare la concessione o la negazione, della relativa autorizzazione».

Tuttavia vorrei aggiungere che non risulta in alcun modo e non è comprovabile che l'accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale dei ministri di Firenze e del tribunale di Livorno (come abbiamo appreso dalla stampa, che ci ha comunicato comunicato l'esito della sentenza, cioè il dispositivo, ma non la motivazione) abbia legittimato quello che potremmo definire l'esautoramento del collegio per i reati ministeriali e delle sue attribuzioni costituzionali Innanzitutto, la Giunta in questo caso ha omesso lo svolgimento di atti istruttori e la stesura di una relazione motivata e ciò in conseguenza del fatto di non aver potuto esaminare nemmeno quegli atti che avrebbero dovuto pervenirle dal tribunale competente. Pronunciarsi su una richiesta che non è mai pervenuta, negando l'autorizzazione a procedere su richiesta dell'interessato e sulla base delle sue argomentazioni, significa porre la decisione parlamentare sulla ministerialità del fatto, *sic et simpliciter*, senza alcuna motivazione, senza alcuna ragionevolezza, sotto lo scudo della valutazione insindacabile di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale. Se tutto questo è vero (e al di là della modestia, se vogliamo, del caso e anche dell'aspetto ridicolo della vicenda, che giustamente ha messo in luce il collega è possibile mai che oggi davvero il Senato voglia assumere una decisione così grave - cioè quella di violare sostanzialmente la Costituzione, violare la legge, violare i Regolamenti -

e possa ripercorrere quella procedura che invece è stata violata? Sempre che, naturalmente, il giudice ordinario o, per meglio dire, il collegio per i reati ministeriali abbia qualche intenzione di investirla. Rimettere esclusivamente alla decisione di un componente del Parlamento la possibilità di stabilire se il fatto che ha commesso è un reato ministeriale è una grave violazione ed è una grave alterazione del principio di ragionevolezza. Ma è anche una violazione - che, a quanto pare, non sembra in questo caso interessare nessuno - del principio della difesa, che invece giustamente è stato richiamato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dal collega Sanna. La procedura è talmente anomala che chi vuole che venga portata a compimento con l'appoggio della maggioranza ritiene che si possano anche violare i suoi diritti, oltre che le prerogative del giudice ordinario. Sotto questo aspetto credo che che tale procedura non possa essere accettata, e vi propongo tre soluzioni finali: o respingere o sospendere, ed attendere il giudizio - cosa che potrebbe essere ragionevole - o rimettere gli atti alla Giunta delle colleghi senatori, ci troviamo oggi di fronte a una procedura ingiustificabile, come hanno detto molti colleghi che mi hanno preceduto, a cominciare dal collega Sanna. Su spinta decisiva della Presidenza del Senato, avallata dalla maggioranza della Giunta, si è operata una forzatura da almeno quattro punti di vista. In primo luogo, si tratta di una forzatura temporale: il caso in questione, che si riferisce al senatore Castelli, è indubbiamente per vari aspetti analogo a quello che ha riguardato l'allora deputato Matteoli. Si tratta infatti dell'ammissibilità di una valutazione pregiudiziale del Parlamento sul carattere ministeriale di un reato. Il punto è che la Corte costituzionale ha recentemente pubblicato il solo dispositivo sul caso Matteoli, ma non ancora le motivazioni, che saranno disponibili a breve. Non si vede perché non si possa attendere tale pubblicazione. In secondo luogo, si tratta di una probabile forzatura in termini di innovazione procedurale, giacché, sempre che ciò non sia consentito dalle motivazioni della sentenza della Corte (che però, per l'appunto, non conosciamo), si considera ammissibile, a differenza di quanto previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dalla conseguente normativa ordinaria, che la Camera di appartenenza valuti la ministerialità di un reato direttamente su richiesta dell'interessato, a prescindere dalla richiesta del competente tribunale dei ministri. Una forzatura che, nonostante la sua assoluta novità, il Presidente del Senato non ha ritenuto di sottoporre all'esame della Giunta per il Regolamento, malgrado l'opportuno invito in tal senso formulato per ben due volte per lettera dal presidente Follini. In terzo luogo, si tratta di una certa forzatura per così dire "cumulativa", nel senso di cumulare in un unico momento due procedure diverse: quella sulla pronuncia parlamentare pregiudiziale sulla ministerialità del reato con quella sulla sussistenza di una delle due scriminanti previste dall'articolo 9, comma 3, della citata legge costituzionale. Se si ammettesse la legittimità della pronuncia parlamentare pregiudiziale bisognerebbe comunque dare la possibilità al tribunale dei ministri di compiere atti istruttori per consentire al Senato di deliberare senza esautorare l'autorità giurisdizionale delle sue attribuzioni costituzionali. Un conto è infatti, ammesso che la Corte lo ritenga legittimo (e per l'appunto ancora non lo sappiamo), avviare la procedura su richiesta dell'interessato, un altro saltare del tutto le competenze dell'autorità giudiziaria nell'istruire la procedura sulla fattispecie di reato. In altri termini, decidendo contestualmente su una pregiudiziale declaratoria della ministerialità del reato e sulla sussistenza dell'esimente, si propone al Senato di pronunciarsi su una richiesta mai pervenuta e soprattutto mai istruita. Si negherebbe l'autorizzazione a procedere su richiesta dell'interessato e sulla sola base delle sue argomentazioni. In quarto luogo, vi è una forzatura in termini di omissione. Resta infatti in ombra l'unica possibile decisione che il Senato potrebbe assumere: il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale in relazione all'ordinanza del 2004 del tribunale dei ministri, formalmente non comunicata al Senato, ed anche nei confronti del giudice penale di Roma per impedire a quest'ultimo di poter proseguire il giudizio penale. Non sono sufficienti quattro gravi forzature a far ritenere che la Presidenza del Senato, in raccordo con la maggioranza della Giunta, abbia violato il proprio ruolo di organo di garanzia, per di più saltando del tutto la Giunta per il Regolamento? Sta venendo meno la lunga tradizione di garanzia della Presidenza del Senato e proprio nel momento in cui ve ne sarebbe più bisogno, in una legislatura in cui la forza dei numeri espone la maggioranza a gravi tentazioni di forzature sulle regole. Non vorremmo essere indotti a pensare che queste nuove procedure per così dire molto innovative e le novità di sostanza a cui potrebbero preludere, che potrebbero consistere in un'interpretazione latissima del concetto di reati ministeriali, in questo, ma soprattutto in altri casi futuri, fossero delle garanzie minori, una sorta di piccolo paracadute d'emergenza in caso di bocciatura da parte della Corte del cosiddetto lodo Alfano. Un qualcosa del genere, sia pure in forma più *soft*, lo aveva prefigurato prima il collega D'Alia, quando diceva che si è partiti dall'abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione e si cerca poi di riparare con vizi di procedure in altro modo. Ma anche senza bisogno di arrivare a questo, appare evidente la logica di scambi di protezione reciproca, tra quella assicurata al Presidente del Consiglio e quella richiesta in cambio per un ex Ministro, con l'avallo della Presidenza dell'Assemblea, la cui registrazione passiva non farebbe certo onore a questo Senato. Per tale motivo bisogna radicalmente opporsi a questo tipo di gravi forzature. Signora Presidente, onorevoli senatori, in una trasmissione denominata "Telecamere" un Ministro della Repubblica disse: «Piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu, preferisco saltare». È da qui e da altre frasi che nasce l'oggetto del procedimento di cui oggi è interessata l'Aula di questo tribunale. Il ben poco onorevole comportamento di personaggi politici che approfittano dell'accesso preferenziale ai che ad essi è consentito più che ad altri, notoriamente - per diffamare ed ingiuriare chi non dispone invece, per difendersi, degli stessi strumenti non è una novità nel nostro Paese. In una coraggiosa sentenza del 1911, mi piace ricordare, il tribunale di Verona ebbe a riconoscere all'offeso il diritto di ritorsione, quasi l'immunità parlamentare si estendesse anche a lui. Un ragionamento che avrebbe perfettamente senso ancora oggi, se è vero che l'istituto dell'immunità è pur sempre ispirato all'esigenza di garantire la libertà della funzione di governo, e non di assicurare un privilegio ai Ministri. Il sistema democratico, dunque, si gioverebbe di un'estensione dell'immunità al privato che, offeso dai giudizi espressi dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, esprimesse a sua volta i suoi giudizi in merito all'accusa e all'accusatore, senza dover dover temere una querela da parte di quest'ultimo. Il dilagare di comportamenti diffamatori da parte di parlamentari eroicamente pronti a nascondersi dietro alla loro insindacabilità ha indotto la Corte costituzionale alla nota evoluzione giurisprudenziale sul nesso funzionale: la *ratio decidendi* ha una forza espansiva che la dottrina unanime ha considerato incontenibile ogniqualvolta - come dice la sentenza stessa la parte lesa vedrebbe altrimenti «compromessa la stessa possibilità (...) di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti». Se la Corte costituzionale, di fronte al caso Castelli, investita dal Senato, dovesse pronunciarsi nel merito, affermando l'immunità del Ministro per ogni sorta di esternazione a cui carattere ed ed educazione lo inducono, non v'è dubbio che i privati non solo si vedrebbero negare il ricorso alla giustizia per difendere i propri diritti personali, ma sarebbero oltretutto gabbati, perché se lo sentirebbero dire solo dopo aver faticosamente percorso tutti i gradi dell'estenuante giudizio. Si potrebbe persino aggiungere che, se l'apertura della Corte nei confronti dell'intervento del terzo può valere per i conflitti in cui venga in questione l'insindacabilità dei parlamentari, vale a molto maggior ragione quando invece entri in gioco la pretesa immunità del Ministro. Ragionando con la stessa logica e la stessa etica del tribunale di Verona del 1911, che ho prima ricordato, al privato danneggiato dall'esternazione ministeriale non potrebbe essere neppure concesso il diritto di ritorsione, cioè di esprimere liberamente e e con altrettanta secchezza il suo giudizio su chi lo ha diffamato. Nessuna difesa dialettica, nessuna difesa processuale. Ma, soprattutto, la domanda spontanea è: ne vale la pena? La questione di diritto della determinazione dei limiti di esercizio del diritto di cronaca e di critica politica è rilevante ai fini dell'applicabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione: invocarla nel processo può essere più utile alla causa del di altri inutili tentativi di fuga dal processo, anzi dai due processi. Il limite della verità, che in base all'antico principio della nostra giurisprudenza vieta non solo l'attribuzione di fatti penalmente rilevanti senza una rigorosa verifica, ma anche valutazioni critiche formulate come ipotesi, prescindendo dal necessario accertamento giudiziario, è già stato interpretato evolutivamente in materia di diritto di cronaca. La Corte di cassazione, in un'ottima sentenza delle sezioni unite penali del 2001, ha riconosciuto che la scriminante

contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da escludere la possibilità di censura da parte dell'intervistatore e da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In effetti, la constatazione che il dovere di controllare l'attendibilità della fonte non vada dilatato al punto da paralizzare la divulgazione delle notizie raccolte aveva già fatto dire, con una sentenza del 1988 della Corte di cassazione, del fatto oggetto della notizia dalla verità della notizia come fatto in sé. Perciò, anche qualora il fatto riferimento sia falso, può ben essere vero e risaputo che lo si racconti, costituendo così un fatto rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 12196 del 2001, ha precisato che «il cronista o il critico deve già nella sua propalazione al lettore dare atto che si tratta non di notizia relativa a un fatto riscontrato, ma che l'unico fatto storico riscontrato è che una è che una determinata notizia circoli pubblicamente», con l'ulteriore specificazione del dovere di riferirne anche le fonti di propalazione. Come il diritto di cronaca, anche quello di critica nell'esercizio dell'attività politica è una manifestazione della libertà di pensiero; esso è anche un'estrinsecazione della libertà di concorrere con metodo democratico alla formazione della politica nazionale. Quel metodo democratico, esplicitato come regola di gestione della politica nell'articolo 49 che non comporta solamente l'attribuzione ad ogni cittadino dei diritti di elettorato attivo e passivo, di costituzione e partecipazione ad associazioni politiche, di interpello delle Camere, ma anche il rispetto di altre regole necessarie al regime democratico. Tra queste vi è quella di garantire alla collettività, attraverso mezzi di informazione di massa, ma anche attraverso la pubblica iniziativa di chi dell'attività politica è partecipe, la conoscenza dei fatti di rilevanza politica. In forza di ciò, l'interprete deve tener conto della particolare rilevanza dell'interesse pubblico e della conseguente minore tutela dell'onore personale. È vero: su questo secondo profilo le reticenze giurisprudenziali sono maggiori, ma l'evoluzione si è oramai riscontrata anche qui se, per una banale lite insorta in un parcheggio di auto, la Corte di cassazione ritiene che non vi sia alcuna carica offensiva in «frasi particolarmente colorite», annullando così una condanna per ingiurie, a sintomo che «la coscienza oramai diffusa, arresasi dinanzi al diffondersi di gratuite volgarità anche attraverso il mezzo televisivo» fa passare oltre certe affermazioni. Trattandosi di condotte strettamente strettamente a ridosso del legittimo esercizio del diritto costituzionale di libertà d'espressione, il riscontro dell'esimente del diritto di critica dipende da una valutazione comparativa degli interessi in gioco. Nella loro dimostrazione processuale i reati di opinione devono poter trascolorare in condotte non sanzionabili. Queste conclusioni, tratte dalla sentenza della Corte di cassazione n. 31037 del 2001, traspongono alla materia della critica politica buona parte della giurisprudenza evolutiva già maturata in materia di diritto di cronaca, riferendovi peraltro le due condizioni maturate in quell'ambito per scriminare la diffamazione, il fatto in questione sia attinente alla vita politica nazionale e locale e rivesta un sufficiente grado di interesse per la collettività (requisito della pertinenza) e che la rappresentazione di quel fatto come probabile o possibile sia ragionevole e derivi dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti (requisito

alla quale i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica politica nel caso di specie risiedevano nel fatto che 1'imputato espressamente dichiarò di parlare, nell'assemblea comunale,

tra il comportamento della persona e il comportamento del soggetto che rivestiva una funzione istituzionale o politica che fosse (in quel caso istituzionale). È questa dunque la strada principale per affrontare la questione della salvaguardia, nel nostro ordinamento, del diritto di critica politica; dimenticarsene significherebbe annettere alle immunità un valore diverso ed ulteriore rispetto alla loro funzione precipua, sovraccaricando l'istituto di contenuti non propri e, peggio, differenziando il personale politico politico in virtù del mero dato dell'appartenenza ad un'Assemblea elettiva parlamentare o, peggio ancora, all'Esecutivo. L'indicazione giurisprudenziale offerta come la più conforme ai valori costituzionali trova conferma anche nell'evoluzione della consolidata giurisprudenza convenzionale europea. L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, infatti, riconosce la libertà d'espressione come uno dei cardini indispensabili per una società democratica al punto di riconoscere detta libertà sia nei confronti delle informazioni che anche delle idee. Nella sentenza Lopez Gomes da Silva contro del 28 settembre 2000, che certamente il relatore conoscerà, si precisò infatti che la garanzia della Convenzione riguarda anche queste ultime, sia quelle «colte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, sia quelle che urtano, sorprendono ed inquietano». La ricerca di un difficile equilibrio è una problematica tutt'altro che sconosciuta anche a Strasburgo. La Corte ha sempre spiegato che le limitazioni alla libertà d'espressione devono essere interpretate in maniera ristretta al fine di non svuotare il valore che la libertà d'espressione riveste all'interno di una società, sebbene proprio nella citata sentenza 28 settembre 2000 la Corte abbia finito per affermare che deve essere riconosciuto

secondo paragrafo, della Convenzione. Sul punto, la Corte stessa ebbe ad affermare che tale necessità implica l'esistenza di un «bisogno sociale imperioso» e che, nonostante sia riconosciuto agli Stati un certo margine d'apprezzamento nel giudicare l'esistenza di un tale bisogno, tale margine va di pari passo con un controllo europeo. Nella giurisprudenza della Corte europea «i limiti della critica accettabile sono più larghi con riferimento ai politici che agiscano nella loro pubblica pubblica veste», perché inevitabilmente e consapevolmente si assoggettano allo scrutinio di parole ed atti esercitato da giornalisti e pubblico. Non si vede allora perché si debbano sottrarre dall'esercizio attivo di questo scrutinio anche gli altri soggetti appartenenti alla parte politica di opposizione. E, difatti, non si è mai posto a livello europeo il problema di sanzioni irrogate dall'ordinamento giuridico ad un politico su iniziativa di altro politico che lamentasse il debordaggio dai limiti del diritto di critica. Una prima indicazione giurisprudenziale oltre alle indicazioni suddette è giunta proprio, rinviando alla giurisprudenza della Corte europea, con il decreto del 26 giugno 2003, con cui il giudice per le indagini preliminari di Milano, dottor Guido Salvini, ha disposto il giudizio per il reato di cui agli articoli 81 e 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale nei confronti del senatore Dell'Utri. Il decreto ha limitato il giudizio a solo due dei quattro fatti oggetto della querela dell'Onorato.

che un magistrato nutre o ha manifestato le proprie convinzioni politiche e che tale circostanza giustifica dubbi sull'imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò è avvenuto, secondo il giudice Salvini, nelle dichiarazioni al «Corriere della Sera» del 6 marzo 2002,

di critica affermare che un magistrato ha consapevolmente commesso abuso di potere esercitando nei confronti di un soggetto in senso sfavorevole le proprie funzioni giurisdizionali in appoggio alla presunta strategia di un partito politico. partito politico. Alla luce di questa disamina, il senatore Castelli si tranquillizzi: ha buone *chances*, da ciò che sappiamo, di vedere applicato l'articolo 21 della Costituzione anche a lui. Non cerchi invece una scappatoia che piega uno strumento diverso (quello ministeriale). Invocare l'esimente dell'interesse pubblico per una disputa politica rischia di consacrare - a favore di chi, provvisoriamente, governa - una predominanza che esclude il contraddittore dalla possibilità di chiedere tutela giurisdizionale. I democratici hanno presente la lezione giovannea che distingue l'errore dall'errante: tutto ci divide dalla figura di Diliberto, con rispetto parlando, ma relegarlo al di fuori dell'ordinamento giuridico è contrario alla nostra visione

tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su questo caso. L'ampia relazione del collega Sarro - che ringrazio anche a nome del mio Gruppo per l'ottimo lavoro svolto - mi esonera dal ricostruire i fatti di questa delicata vicenda, che risale al marzo del 2004. 2004. La relazione dimostra inequivocabilmente come il procedimento penale, attualmente pendente dinanzi al tribunale di Roma, nei confronti del senatore Castelli in relazione ad affermazioni chiaramente correlate alla sua attività di Ministro della giustizia sia stato caratterizzato e preceduto da anomalie e ambiguità derivanti da una non corretta applicazione della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, di attuazione dell'articolo 96 della Costituzione, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria. Se c'è un'abnormità, collega Sanna, dobbiamo individuarla nel comportamento della magistratura ordinaria. Dico subito, infatti, che questo caso non avrebbe mai dovuto essere sottoposto alla nostra attenzione. La notizia di reato (mi riferisco alla denuncia-querela per diffamazione presentata dall'onorevole Diliberto in data 27 aprile 2004 nei confronti del senatore Castelli) rappresenta una vera e propria pseudo notizia di reato, da cestinare immediatamente in quanto infondata *ictu oculi*, trattandosi di una querela per frasi pronunciate dal ministro Castelli nel corso di una trasmissione televisiva, da ritenere sicuramente espressione del diritto di critica politica. Poc'anzi il senatore Lusi ha fatto un trattato interessante sul diritto di critica politica;

ad alcuni senatori del mio movimento (in questo caso, al senatore Castelli e poi, vedremo, anche al senatore Divina e a tante altre situazioni). Parte della magistratura ordinaria applica la regola dei due pesi e delle due misure; talvolta verrebbe davvero voglia di parlare di una vera e propria persecuzione politica attuata in forme giudiziarie. Se, infatti, sul cosiddetto caso Petruccioli (recentemente conclusosi con l'assoluzione dell'ex Presidente della Commissione di vigilanza RAI),

96. Il tribunale dei ministri, tuttavia, ha declinato la propria competenza, qualificando diversamente il fatto come reato comune, derubricando l'illecito ascritto al Ministro a semplice reato comune. Nell'assumere tale decisione, il tribunale dei ministri ha posto in essere un procedimento assolutamente atipico, rimettendo gli atti al giudice ordinario senza pronunciare alcun provvedimento di archiviazione, il quale è stato quale è stato comunicato alla Giunta - su nostra richiesta - dopo cinque anni. In forza dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, al Collegio per i reati ministeriali, il tribunale dei ministri, spetta un'alternativa tra due sole opzioni: la trasmissione del decreto di archiviazione al Senato o la richiesta dell'autorizzazione a procedere. Non è ammissibile, da parte del tribunale dei ministri, una semplice declaratoria di incompetenza funzionale (così come è avvenuto nel nostro caso) che, qualificando i fatti come reato comune e non ministeriale, spogli il Senato di ogni possibilità di pronunciarsi. Nel nostro caso non ha trovato attuazione l'articolo 8, comma 4, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989, e ne è derivata una menomazione di quel principio di leale collaborazione che dovrebbe sempre caratterizzare i rapporti tra il Parlamento e l'autorità giudiziaria ordinaria, che ci ha impedito fino ad oggi di esprimere una valutazione in ordine alla sussistenza dei parametri politici, la quale compete unicamente a noi. Questa violazione ha comportato un grave *vulnus* per le nostre prerogative il Senato non ha potuto conoscere tempestivamente la volontà del Collegio per i reati ministeriali. Ci è stata negata la facoltà di esercitare un potere a noi riconosciuto dall'articolo 96 e di dichiarare se sussistano in questo caso i parametri del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, valutazione che il Senato deve compiere nell'ambito delle proprie competenze politiche in un momento anteriore all'esercizio della funzione assegnata alla giurisdizione ordinaria. Siamo sicuramente di fronte ad un reato ministeriale (non credo che nessuno abbia il coraggio di negarlo) e la nozione ampia di reato ministeriale, che ormai tutta la giurisprudenza e la dottrina riconoscono, si attaglia perfettamente alla nostra fattispecie. Dobbiamo ora verificare ed individuare - la relazione del collega Sarro individua perfettamente questo aspetto - quale ipotesi giustificativa della condotta del Ministro possa essere riconosciuta nel nostro caso. Ebbene, onorevoli colleghi, il ministro della giustizia Castelli pronuncia quelle frasi nell'ambito di una trasmissione televisiva dove si discute di lotta al terrorismo e lo fa per contrastare la censura politica dell'ex Ministro della giustizia sull'operato del Governo in materia di giustizia. più chiara di così: il contesto è chiaro e la finalità politica di quelle parole è molto chiara. Ovviamente si tratta di due personalità forti, che hanno caratteri forti, e nell'ambito di un acceso dibattito televisivo ci può stare anche qualche frase che va oltre il limite, ma che - ripeto - ha una connotazione puramente politica. Il fine politico perseguito dal ministro Castelli in quel momento era di tutelare l'immagine di un Governo e di un Dicastero che aveva fatto della lotta al terrorismo il suo obiettivo principale. si potrebbe parlare, anziché di reato ministeriale, di «reato di governo», parafrasando una dottrina che ha scritto saggi importanti sulla responsabilità penale ministeriale. Era davvero una condotta perfettamente ascrivibile alla funzione di governo. Spetta a noi, oggi, valutare comparativamente, in chiave di bilanciamento tra l'interesse leso dal reato di diffamazione e quello perseguito dal ministro Castelli. La condotta del Ministro è stata strumentale al compimento dei doveri legati alla sua carica di Ministro ed è proprio al perseguimento dell'obiettivo della continuità dell'azione ministeriale nella lotta al terrorismo che la Giunta, nella sua relazione, ha attribuito il valore di preminente interesse pubblico.

Signor Presidente, intervengo per motivare la necessità di accogliere gli ordini del giorno che sono stati presentati dal mio Gruppo. Mi consentiranno i colleghi di non tornare approfonditamente sul merito della vicenda che, mi si lasci dire, rispetto alla qualità della questione istituzionale, costituzionale e politica che stiamo affrontando, è poca cosa. Mi permetto sommessamente soltanto di segnalare che nella relazione del senatore Sarro, che ha svolto con molta diligenza il proprio ufficio di relatore, c'è qualche salto logico (mi scuso per il gioco di parole). paradossalmente, appare che la riconducibilità della condotta del ministro Castelli all'esercizio delle funzioni tipiche dei ministri (e, quindi, nel compimento di atti definiti funzionali rispetto alla carica ricoperta) siano così qualificabili per la ragione che il Ministro stesso, mentre offendeva il collega avversario con il quale dibatteva, in realtà lo faceva per essere stato esso stesso attaccato per comportamenti non consoni all'esercizio della funzione ministeriale. Questo è chiaramente un salto logico (un salto logico per proiezione dell'argomento), e vale soltanto a colorare la vicenda di cui ci stiamo occupando di una ulteriore confusione dei termini e delle questioni. Il mio intervento è finalizzato, infatti, esclusivamente a informare quest'Aula, peraltro assai poco frequentata da parte della maggioranza, di quanto sta avvenendo con il voto che ci viene proposto. Non so quanti di voi ricordano che la disciplina del 1989, che modificava l'articolo 96 della Costituzione, è intervenuta per abrogare la norma che attribuiva l'accertamento dei reati ministeriali alla Corte costituzionale e, quindi, per eliminare la preventiva deliberazione parlamentare della messa in stato di accusa. Si attribuiva, quindi, la competenza sui reati ministeriali alla magistratura ordinaria. Era il 1989 e ricordiamo tutti il momento in cui questa decisione maturò. Era ancora viva, vivissima, l'eco del famoso scandalo per le carceri d'oro e, comunque il Parlamento si orientò in maniera quasi unanime

i reati ministeriali venissero sottratti al foro privilegiato della Corte costituzionale e alla preventiva deliberazione parlamentare di messa in stato di accusa e perché i ministri venissero giudicati dalla magistratura ordinaria. Ovviamente, questa riforma prevedeva una fase parlamentare, che ha una funzione di filtro rispetto all'esercizio dell'azione penale e che si innesta dopo che il tribunale dei ministri ha esperito gli accertamenti preliminari e ha ritenuto già la natura ministeriale del reato. Che sia chiaro: non è reato ministeriale solo quello che viene commesso da chi è ministro nel periodo di tempo in cui accade il fatto, il fatto, ma, secondo la lettera dell'articolo 96 della Costituzione, il reato commesso nell'esercizio della funzione ministeriale. È chiaro, quindi, cosa facemmo nel 1989! Nell'eventuale fase parlamentare, poi, le Camere possono negare l'autorizzazione in due casi specifici: quando l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o quando abbia perseguito un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Perdonatemi, ma nella relazione del senatore Sarro, a un certo punto, si dice che il ministro Castelli avrebbe agito per

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, che ha attuato la riforma costituzionale, stabilisce che il tribunale dei ministri deve disporre l'archiviazione, tra i vari casi, quando ritenga che il fatto integra un reato diverso da quelli indicati dall'articolo 96 della Costituzione. Quindi, non quando rileva che il soggetto inquisito era ministro della Repubblica. Si deve invece trattare di un reato connesso all'esercizio della funzione La categoria del reato ministeriale, secondo la dottrina e la giurisprudenza più recente, riguarda la competenza funzionale del soggetto, quindi la particolare qualificazione soggettiva dell'autore ed il rapporto di connessione tra la condotta e le funzioni esercitate dal ministro. Credo che su questo non possano esserci dubbi. Per scrupolo sono andata a riguardarmi tutti gli atti parlamentari di Camera e Senato. Andateveli a rileggere e vedrete qual era la nostra volontà, al di là delle persone fisiche; io c'ero, ma non è questo il punto. punto. Cosa stiamo facendo, se accogliamo la proposta della Giunta? Di fatto modifichiamo l'articolo 96 della Costituzione, così come riformato nel 1989, la sua *ratio*, la sua finalità ed i suoi limiti. Il Senato non è senza strumenti. Il Parlamento non è senza strumenti. Noi lo sappiamo benissimo, perché ne abbiamo esperienza. Quando una pronuncia del tribunale dei ministri

da parte del tribunale dei ministri non ha avvertito il Senato. Ma proprio questa è la questione che pende davanti alla Corte, esattamente questa, che secondo me può essere risolta, anche in via interpretativa. Infatti,

del competente tribunale dei ministri, la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica e il dovere di quest'ultimo di trasmettere quell'archiviazione al Senato. Questo passaggio manca, ma la soluzione è già nella legge e comunque è su questo punto che quella famosa sentenza della Corte costituzionale che dovremmo attendere interviene. Ma al posto del conflitto di attribuzione, noi stabiliamo invece un principio abnorme - come è stato detto qui - fuori da ogni regola, fuori dall'ordinamento,

e investe la Giunta, che comincia a maneggiare aspetti delicatissimi come quelli che riguardano, appunto, le attribuzioni previste dalla Costituzione e dalla legge costituzionale in materia. Quindi, un potere abnorme, esercitato in maniera abnorme, scansando il risultato, l'esito, dalla sede propria, che è quella del conflitto di attribuzione, addirittura dicendo che si è dicendo che si è abilitati a riconoscere la presenza, nel fatto contestato, dell'esimente del perseguimento da parte del ministro dell'interesse pubblico preminente. Cosa sta accadendo sta accadendo allora? Con la prassi che instauriamo, con questa decisione di oggi, non solo travolgiamo un sistema che è fatto dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge n. 219, ma facciamo di più, cari colleghi. Stiamo introducendo un'immunità ministeriale che non è prevista da nessuna parte e che la riforma del 1989 intendeva eliminare; andiamo contro un deliberato del più alto rango, quello costituzionale, adottato dal Parlamento; stabiliamo l'immunità *on call* richiesta dai ministri e la affidiamo alle maggioranze parlamentari. Questo è ovviamente il risultato che volevate raggiungere, ossia completare, per la parte in cui non siete riusciti, l'usbergo del lodo Alfano estendendolo ai Ministri richiesta che ha la forza di dire «tu sì e io no», una richiesta che è politica e sta sconvolgendo il nostro quadro costituzionale.

la legge costituzionale e un sistema di equilibrio delicatissimo che riguarda la relazione tra il Parlamento, il Consiglio dei ministri e i suoi componenti e la giurisdizione ordinaria.

Dichiaro chiusa la discussione. Avverto che da parte del prescritto numero di senatori sono stati presentati gli ordini del giorno

Grazie, Presidente.

solleva aspetti giuridici che non solo hanno occasionato precedentemente pronunce da parte del tribunale dei ministri e della Corte costituzionale, ma anche la necessità da parte della Giunta di svolgere un'azione approfondita e sostanzialmente sostanzialmente integratrice, cercando di ripristinare una fattispecie procedimentale che in questa vicenda è stata completamente alterata, certamente non per responsabilità del Parlamento, ma per negligenze o inadempienze dell'autorità giudiziaria. Nella mia brevissima replica e nel tentativo di confutare molte delle obiezioni e dei rilievi che sono stati mossi, partire dall'ultimo intervento, quello della senatrice Finocchiaro, a proposito dell'impianto che nel nostro ordinamento, dopo la revisione dell'articolo 96 della il procedimento per il riconoscimento della ministerialità dei reati. Effettivamente, la riforma dell'articolo 96 si è mossa in quella direzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 e la successiva legge ordinaria di attuazione, la n. hanno delineato un meccanismo abbastanza chiaro. Il procedimento comprende una prima fase rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, una seconda fase propria del Parlamento e una terza fase, eventuale, che è nuovamente dell'autorità giudiziaria e che segna, dopo l'esaurimento della fase parlamentare, l'avvio delle indagini che in senso tecnico si

La legge costituzionale individua con precisione gli atti che formalmente segnano l'inizio e la conclusione di questa fase. L'atto d'inizio è la ricezione da parte del procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto della corte d'appello competente per territorio della *notizia criminis* e la trasmissione al collegio ministeriale, come precisa la legge costituzionale senza condurre alcuna indagine; l'atto conclusivo è quello con cui, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n.1 del 1989, lo stesso procuratore della Repubblica rimette alla Camera di appartenenza del Ministro oggetto del procedimento le conclusioni e dunque l'atto finale della verifica preventiva. Nel nostro caso sono questi gli atti che sono mancati e che poi hanno alterato la corretta sequenza procedimentale. È in ragione di questo fatto che la Giunta, con una nota del suo Presidente Presidente che recepiva l'indirizzo e il dibattito espresso tanto in Giunta quanto nell'Ufficio di Presidenza, ha chiesto al Presidente del Senato che che si acquisisse dapprima l'ordinanza del tribunale dei ministri e solo successivamente il provvedimento di comunicazione con il quale il procuratore della Repubblica competente indica quali sono le conclusioni e le valutazioni finali di questa fase preventiva, preliminare. È dunque a partire da quel momento che

della prima fase, vale a dire tanto che si arrivi ad un'archiviazione quanto che si arrivi ad una declaratoria del difetto di ministerialità del reato e quindi si renda necessaria una prosecuzione ordinaria del procedimento. D'altra parte, questa conclusione è avvalorata dalla interpretazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, che da questo punto di vista, vista, applicando le regole ermeneutiche correnti, ordinarie, i principi fissati dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, è chiarissima.

ovvero che il fatto in contestazione non sia riconducibile nell'ambito della previsione dell'articolo 96 della Costituzione, e quindi non sia riscontrabile il carattere ministeriale del reato, dispone l'archiviazione. Allora se un rilievo critico va mosso, è all'uso di questo termine che genera facilmente confusione o comunque la tendenza ad immaginare il provvedimento di archiviazione così come disciplinato dalle norme del codice di procedura penale. In realtà, è il provvedimento di chiusura di quella fase, che va trasmesso al Parlamento e che va accompagnato,

caso recede anche la posizione della lettera del senatore Castelli, che non è un atto di impulso o che ha dato avvio al procedimento. Il procedimento ha avuto inizio con la prima comunicazione fatta dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma e rimessa al Senato, che ha seguito un suo *iter*. La posizione e la lettera del senatore Castelli hanno avuto esclusivamente una funzione di sollecito per la ripresa del procedimento e per l'avvio della fase parlamentare obbligatoriamente prevista. prevista. Ciò, naturalmente, supera anche il rilievo mosso dal senatore Li Gotti a proposito del precedente costituito dalla lettera della Presidenza del Senato del gennaio 2006, essendo la questione (cui quella lettera e la determinazione facevano riferimento) fondata su presupposti di fatto completamente differenti. Infatti, in quel caso, la richiesta di attivazione del procedimento avveniva in assenza di qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel nostro caso la fase di valutazione preventiva di competenza dell'autorità giudiziaria si era materializzata: non era del tutto perfezionata perché mancava l'atto di comunicazione finale, ma la pronuncia esisteva

su richiesta del senatore Castelli, ma riprende dopo che, a seguito dell'attività istruttoria della Giunta, la fase preliminare si è chiusa e si passa alla fase parlamentare. Sempre in replica alle osservazioni del senatore Li Gotti che, con la sua consueta suggestione dialettica, ripropone un argomento che ha già posto anche in Giunta a proposito della ministerialità del reato,

la qualificazione in termini di ingiuria delle affermazioni fatte dal senatore Castelli nel corso della trasmissione, che riguardano aspetti strettamente attinenti all'attività di governo e profili

era riferita alla qualificazione dell'interesse specifico in aggiunta all'interesse generale, normalmente tutelati nel nostro ordinamento da un provvedimento legislativo e garantiti dall'azione di governo. Ovviamente, la difesa di un provvedimento legislativo - nel caso specifico, le misure per la lotta al terrorismo e la riforma dell'ordinamento giudiziario - e dell'azione di governo su queste tematiche rappresentano un'affermazione politicamente impegnativa,

oggetto di protezione dell'atto legislativo difeso dal senatore Castelli ad avere una rilevanza, proprio perché interessi attinenti alle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione. Mi avvio a concludere la replica,

Dobbiamo considerare che in questa vicenda abbiamo una pronuncia della Corte costituzionale che ricostruisce autorevolmente e puntualmente tutti gli accadimenti,

e l'attività della Giunta delle immunità che, nella XIV legislatura, esaminando questo caso specifico, ha audito il senatore Castelli. Abbiamo, quindi, un insieme copioso e significativo di elementi che hanno permesso alla Giunta di condurre la sua valutazione,

Pertanto, non c'era, né è stata ravvisata l'esigenza di condurre alcun espletamento istruttorio, né tantomeno sono state menomate le prerogative di difesa del senatore Castelli, atteso che le sue ragioni, proprio sulla qualificazione di quei fatti, erano contenute nella lettera inviata al Senato e quindi alla Giunta per l'esame successivo. all'intervento del senatore Lusi, certamente sulla questione complessa ed articolata della tutela del diritto del terzo nel giudizio per il conflitto di attribuzione è un tema importantissimo ma *de iure condendo*. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 21 alle affermazioni del senatore Castelli, in questo caso non ci si sottrae alla valutazione del giudizio ordinario, temendo quello che può essere l'esito, perché è un aspetto che non interessa né la Giunta né l'Assemblea. Qui si discute di quelle che sono le prerogative del Parlamento e la loro difesa, che in questo loro difesa, che in questo caso sono state seriamente compromesse da un'azione non esaustiva e soprattutto non rispettosa delle disposizioni sul procedimento e sugli adempimenti che andavano fatti e che hanno generato una situazione complessa, complessa, per certi versi anche confusa, che la Giunta col suo lavoro ha cercato di ripristinare nella sua corretta successione, rassegnando oggi le conclusioni che nella relazione introduttiva sono state indicate.

di attendere qualche giorno la motivazione della Corte costituzionale sulla interpretazione che deve darsi ad alcune normative specifiche che riguardano anche il nostro caso, ritenendo che proprio questa discussione abbia evidenziato la difficoltà di trovare una soluzione. Sperando di coglierci, speriamo oggi di decidere negli stessi termini in cui la Corte costituzionale ha già deciso, ma non ha ancora scritto, o di cui comunque non esiste ancora la motivazione. In una materia motivazione. In una materia così delicata non si può sperare: bisogna decidere con convinzione e con chiarezza di valutazione. Allora ritenere opportuno, proprio all'esito di questa discussione, di consentire un accrescimento delle nostre conoscenze ed un orientamento certo in materia di norme costituzionali

formulata, la Giunta ha richiesto un voto cumulativo su due diverse questioni. Si chiede di votare

dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Sono due pronunce che avvengono in un unico contesto. Non so se sia o meno opportuno procedere eventualmente ad un voto disgiunto, perché si tratta di due materie diverse. Una volta acquisito il voto sulla ministerialità o meno, si può passare alla seconda votazione.

comunque ancorato a ciò che è stato detto nel corso della discussione generale, nonostante - me ne rendo conto - gli sforzi giuridici compiuti dal relatore Sarro,

Relatore Sarro e colleghi del Senato, ciò che stiamo affrontando non è una disquisizione sull'ordinamento giudiziario e sulla lotta alla criminalità organizzata.

o censurato il senatore Castelli di avere saltellato gridando: «Chi non salta, italiano è»; il senatore Castelli gli «Piuttosto che mandare in giro a sprangare, come fai tu, preferisco saltare». Ciò che veniva difeso in quel momento dal senatore Castelli era il saltare, non l'ordinamento giudiziario o la normativa antimafia. Egli ha cioè risposto a Diliberto rivendicando la legittimità

Mi sembra proprio che non possa ritenersi convincente la tesi per cui il saltellare sia un atto ministeriale: sarà un'altra cosa, utile anche al fisico, ma non è un atto ministeriale. Ecco perché voteremo no alla proposta della Giunta.

il modo civile e pacato, ma anche approfondito, con cui il collega Sarro ha risposto alle obiezioni emerse nel corso del dibattito. Ci sembra però che nel corso del dibattito, soprattutto alla fine, alcuni interventi abbiano esageratamente alzato il tono politico.

intendesse tendenzialmente limitare l'intervento parlamentare nel fissare i reati ministeriali;

Il senatore Casson si riferiva alla necessità di attendere le motivazioni di una sentenza della Corte costituzionale, della quale abbiamo letto una decina di giorni fa sui giornali, in un caso per certi versi analogo e per altri molto diverso, in ordine al quale i giornali hanno scritto che la Corte costituzionale, contraddicendo la proposta del relatore, professor De Siervo, ha stabilito il principio che sia il Parlamento a fissare la ministerialità dei reati.

il lodo Alfano, la Corte costituzionale e altre vicende che vogliamo mantenere distinte.

il punto politico, anzi, se me lo consentite, di politica costituzionale è che la giurisdizione non può essere una macchina da guerra senza ambiti e senza limiti. Gli ambiti e i limiti della giurisdizione li fissa la Costituzione. È la Costituzione che si scrive sempre con la lettera maiuscola, non la giurisdizione.

ci ricorda che a quella trasmissione televisiva erano invitati anche l'onorevole Diliberto, guarda caso ex Ministro, il presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Gaetano Pecorella, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Edmondo Bruti Liberati. Mi sembra che si possa dedurre che il senatore Castelli non era stato invitato

È allora lecito in questa occasione domandarsi perché mai la libertà di parola, in quel tipo di trasmissione televisiva, non debba essere la stessa di un Ministro quando parla in Parlamento. La Costituzione è fatta di cose complesse, è complicata, ma è fatta anche di valori semplici e nitidi. Ricordo - lo vidi in televisione, non ero senatore - con quanta sofferenza interiore l'allora presidente del Senato Marini non volle minimamente scalfire la libertà di parola di un Ministro (mi pare fosse Padoa-Schioppa) che in quest'Aula ricorreva anche ad insulti (fra virgolette) di carattere personale nei confronti di un generale per illustrare una posizione politica. Ecco, proprio in nome di quella libertà di parola noi riteniamo che la Giunta abbia fatto bene a non tenere sulla graticola ancora a lungo il senatore Castelli. È per tutti questi argomenti - che volutamente non abbiamo allargato al dibattito politico - che votiamo a favore delle conclusioni della Giunta, sperando di far bene, nell'interesse di un più civile e pacato rapporto fra la giurisdizione, con la minuscola, e la Costituzione, sempre con la maiuscola.

dicevo, sono stati presentati tre ordini del giorno, ma la Presidenza ritiene che l'eventuale

Ricordo che in applicazione analogica dell'articolo 135-*bis*, comma 8, ultimo periodo, la proposta della Giunta si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Altresì, in applicazione analogica dell'articolo 135-*bis*, comma 8-*bis*, del Regolamento, il risultato della votazione nominale con procedimento elettronico che ora effettueremo non sarà immediatamente proclamato in quanto i senatori che non abbiano partecipato al voto potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari, che ne prenderanno nota in apposito verbale,

Ricordo nuovamente che i senatori che non abbiano partecipato alla votazione elettronica potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari che ne prenderanno nota negli appositi verbali, nel corso di questa seduta e della seduta pomeridiana di oggi, sino alle ore 19. Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno,

per i disegni di legge: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009"

Presidente, onorevoli senatori, le principali novità relative all'esercizio finanziario 2008 concernenti il conto del bilancio si riscontrano nella nuova struttura di classificazione del bilancio dello Stato, articolato su due livelli di aggregazione: missioni e programmi. Questa articolazione, già avviata in fase sperimentale nel 2007, tende a garantire una migliore informazione sull'insieme complessivo delle risorse disponibili per il perseguimento di specifiche finalità pubbliche. Il conto consuntivo finanziario per l'anno 2008 è costruito pertanto, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base delle missioni, che sono realizzate attraverso uno o più programmi. Questi ultimi sono, a loro volta, suddivisi in macroaggregati (le nuove UPB), i quali sono articolati, nell'ambito di ciascun centro di responsabilità amministrativa, in capitoli, così da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in riferimento agli obiettivi previsti. Tale nuova classificazione funzionale del bilancio rappresenta una innovazione che ha riscosso giudizi positivi in più sedi, in quanto concentra l'attenzione sulle finalità e sui risultati dell'azione amministrativa. Da ciò dovrebbe conseguire in prospettiva una valorizzazione del ruolo del rendiconto, che diventa la sede della valutazione delle politiche pubbliche, costituendo il documento contabile che consente, da un lato, di dar conto *a posteriori* dei risultati della gestione da parte del Governo nei confronti del Parlamento e, dall'altro, di tener conto dei risultati della gestione in vista dei processi di autocorrezione e di effettuazione delle nuove scelte. Le proposte sono articolate per ciascun esercizio del bilancio pluriennale, conferendo maggiore certezza alla pianificazione delle attività. L'ampliamento dell'orizzonte temporale del bilancio da uno a tre anni, infatti, comporta una proiezione triennale completa, definendo la manovra necessaria per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun esercizio; in precedenza, le manovre hanno operato la correzione per il primo anno, mentre la proiezione triennale avvicinava il saldo di ciascuno degli esercizi successivi all'obiettivo programmatico. Va detto, per completezza, che sul punto permangono comunque talune criticità, quali le incongruenze nella ripartizione a livello di missioni e difficoltà nei rapporti tra articolazioni organizzative e nuove aggregazioni, specie se comuni a più centri di responsabilità amministrativa. Si tratta comunque di aspetti suscettibili di soluzione non complessa. A seguito della nuova classificazione del bilancio, le note preliminari di consuntivo a corredo del conto consuntivo delle Amministrazioni dello Stato, previste dall'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, presentano una nuova stesura con lo scopo di illustrare i risultati conseguiti dai Ministeri in relazione agli indirizzi del programma di Governo, avvalendosi anche degli indicatori individuati inizialmente. Venendo ai dati dell'esercizio, va rammentato che il rendiconto generale dello Stato rappresenta la sede formale in cui il Parlamento esercita la funzione costituzionale di verifica degli elementi finanziari del bilancio annuale. In via preliminare, si conferma il divario tra i dati di previsione e i risultati di gestione di competenza delle entrate e delle spese; un elemento in qualche misura fisiologico, che tuttavia evidenzia, anche per il 2008, una sensibile differenza nel confronto dei dati consuntivi con le previsioni definitive e con quelle iniziali. Nel raffronto dei dati concernenti le previsioni di entrate e spese iniziali con quelle definitive, nel complesso, le previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali sono cresciute dello 0,2 per cento contro un incremento del 3,7 per cento registrato nel 2007.

L'incremento manifestatosi rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente all'aumento dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 14,9 per cento, mentre sostanzialmente stabili sono rimaste le entrate tributarie ed extratributarie.

Tale andamento è il risultato di una riduzione del 5 per cento dei consumi intermedi, della restituzione e del rimborso di imposte dirette e indirette del 5,6 per cento, rispetto al passato esercizio, di un incremento di trasferimenti correnti alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali del 7,5

Rispetto al passato esercizio, le spese complessive in termini previsionali sono aumentate del 6,4 per cento. Un ulteriore elemento da sottolineare è relativo all'andamento dei saldi di competenza del conto del bilancio. Il saldo netto da impiegare risulta pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a meno 37.991 milioni di euro, e quindi in sensibile regresso rispetto al 2007, Inoltre, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, il saldo assume un valore pari a meno 30.507 milioni, a fronte del dato di 12.406 milioni di euro segnato nel 2007. Occorre comunque osservare che il valore del saldo risulta rientrare nel limite massimo di 34.000 milioni di euro fissato dalla legge finanziaria per il 2008. Evidenzia anche un ulteriore peggioramento del dato relativo all'avanzo primario,

Il ricorso al mercato si è a sua volta attestato a 222.798 milioni di euro (era stato di 154.874 milioni di euro nel 2007, allorché si era evidenziato già un aumento di 4.203 milioni rispetto al 2006). Anche il valore del ricorso al mercato risulta peraltro inferiore al limite massimo, pari a 245.000 milioni di euro (240.500 milioni di euro nel 2007), fissato dalla legge finanziaria per il 2008. Il saldo corrente, il cosiddetto risparmio pubblico, nel 2008 è risultato pari a 22.880 (nel 2007 era stato pari a 56.361 milioni di euro), risultando in netta flessione rispetto al 2007, allorché era invece risultato superiore rispetto all'anno 2006 in cui era stato di 49.983 milioni di euro. Come ha segnalato anche la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto, dai saldi di bilancio si evince come il 2008 sia stato per i conti pubblici un anno decisamente meno positivo del precedente, nel quale si sono esplicati gli effetti di un contesto economico, gravato da una forte recessione internazionale. A margine, avuto riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è salito a 43 miliardi di euro, il doppio rispetto al In percentuale del prodotto interno lordo, si è passati dall'1,5 al 2,7 per cento. Il saldo strutturale - depurato cioè dagli effetti del ciclo economico e dal complesso delle misure *una tantum* - è passato dal 2,9 al 3,4 per Del pari deteriorato è il rapporto debito/PIL che ha invertito la tendenza, tornando ad aumentare rapidamente dal 103,5 per cento del 2007 al 105,7. La crescita nominale dello *stock* di debito pubblico è stata di 63,6 miliardi (contro 17,0 miliardi del 2007), importo determinato, oltre che dal nuovo fabbisogno dell'anno (48,3 miliardi), dall'aumento delle disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia

di competenza, l'entità complessiva degli accertamenti in entrata, incluse le entrate per accensione prestiti, è risultata pari a 720.236 milioni di euro,

In particolare, le entrate finali sono aumentate di 1.925 milioni rispetto al 2007 a fronte di un marcato aumento delle spese finali di circa 45.391 milioni di euro, pari a più 9,2 Dal lato dell'entrata, in particolare, evidenzia, rispetto alle previsioni definitive, un'evoluzione riduttiva degli accertamenti del settore tributario per 7.416 milioni di euro, i cui accertamenti raggiungono 446.165 milioni di euro (solo più 0,5 per cento rispetto al 2007) Sul versante della spesa, la gestione ha dato luogo ad impegni complessivi per 720.544 milioni che riguardano le operazioni finali per 535.737 milioni di euro e le operazioni di rimborso di passività finanziarie per 184.808 milioni di euro. Nell'ambito delle uscite correnti, in particolare, il comparto delle spese di funzionamento ha registrato impegni per 91.053 milioni, quello per interventi per 282.152 milioni, quello degli oneri comuni per 19.058 milioni e quello per gli oneri del debito pubblico per 80.423 milioni di euro, Nel complesso, osserva che il 2008 registra un sensibile deterioramento degli equilibri finanziari dal momento che, a fronte di un solo lieve incremento delle entrate, tale esercizio vede accompagnarsi un significativo aumento delle spese. Il conto dei residui, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2008 e quindi in relazione alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti, presenta un'eccedenza attiva pari a 51.836 milioni, come saldo tra residui attivi per

ringraziando il Presidente e i membri della Commissione bilancio, unitamente al Governo, per il lavoro svolto e gli Uffici per la collaborazione, desidero porre all'attenzione dell'Aula alcuni interessanti contributi formulati dalle altre Commissioni nell'esame del disegno di legge in sede consultiva. In particolare vorrei richiamare il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, dove si rileva che l'esercizio 2008 fa registrare, per la prima volta dopo molti anni, l'arresto del progressivo aumento della quota di residui considerati non esigibili,

che l'effettiva acquisizione in bilancio di tali somme non è affatto scontata. Le incongrue modalità di quantificazione degli accertamenti comportano una loro sistematica sovrastima, che si protrae nel tempo nonostante i rimedi normativamente previsti per la riduzione dei crediti in relazione al loro grado di esigibilità. La Commissione igiene e sanità ha rilevato poi l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione all'adeguatezza della spesa sanitaria, auspicando che siano individuati per il futuro degli indicatori quanto più rigorosi e raccomandando una compilazione più puntuale delle schede di verifica sugli obiettivi. La risposta puntuale a questa esigenza sarà senz'altro data con l'attuazione della legge sul federalismo fiscale che deve essere quindi sostenuta. Va infine ricordato - secondo quanto riportato nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea - che il rendiconto si riferisce ad un anno in cui l'economia mondiale è entrata in una fase di profonda recessione

l'andamento del deficit, nonostante l'esplodere della crisi, non ha portato allo sforamento della soglia del 3 per cento, a differenza dei disavanzi registrati da altri grandi Paesi come Francia, Regno Unito e Spagna, e che, con l'anticipazione all'estate della manovra correttiva di bilancio, l'Italia ha potuto affrontare la recessione con misure di contenimento del disavanzo già incorporate nella legislazione vigente. [**VOTAZIONI

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'anno in corso la crisi economico-finanziaria ha provocato una forte decelerazione dell'economia internazionale e una inversione pressoché generalizzata del prodotto interno dei maggiori Paesi industrializzati. In questo contesto, l'azione di politica economica ha dovuto contemperare l'esigenza di implementare misure antirecessive con la presenza di un elevato debito pubblico e la necessità di evitare effetti negativi connessi ad un potenziale aumento dei tassi di interesse sul debito stesso. Il Governo ha cercato di massimizzare l'efficacia degli interventi nonostante la presenza di forti vincoli di bilancio. Gli interventi sono stati realizzati in modo tale da risultare quanto più possibile neutrali in termini di saldo di bilancio. Tale impostazione è risultata necessaria per l'alto livello del debito pubblico in relazione al prodotto interno, rapporto che è destinato ad accrescersi nel biennio 2009-2010 per effetto del peggioramento del disavanzo pubblico dovuto principalmente all'operare degli stabilizzatori automatici. Nello specifico, il disegno di legge di assestamento al nostro esame contiene, come di consueto, l'aggiornamento, a metà esercizio, delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge e si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio trascorso, dal quale risulta l'entità effettiva dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio finanziario in corso. I dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2009 evidenziano un peggioramento dei saldi di bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2009. Si tratta dell'ovvio effetto del peggioramento delle prospettive economiche connesso alla crisi internazionale. Anzitutto, per quanto riguarda la competenza, il saldo netto da finanziare passa da 32.790 milioni a 69.659 milioni, con un peggioramento di 36.869 milioni; il risparmio pubblico, che nelle previsioni iniziali aveva un valore positivo di 12.748 milioni, milioni, registra un peggioramento di 32.356 milioni ed espone un valore negativo di 19.608 milioni. Il ricorso al mercato, infine, denota un incremento da 255.105 milioni a 292.023 milioni, con un peggioramento di 36.918 milioni; analogo significativo peggioramento si riscontra anche con riferimento all'avanzo primario, che passa da 48.530 milioni a 8.514 milioni, con un decremento di 40.016 milioni. Tali variazioni risultano dalla contrazione delle entrate finali per 26.200 milioni e dal contestuale aumento delle spese finali per 10.670 milioni. Le minori entrate derivano da una diminuzione relativa al comparto tributario pari a 29.379 milioni, solo in piccola parte compensata dall'aumento delle entrate extratributarie per 2.952 milioni e di quelle del titolo III per 228 milioni. Le maggiori spese, pari a 10.670 milioni, derivano da un aumento degli oneri di natura corrente, al netto degli interessi, per un ammontare di 9.076 milioni e dall'incremento delle spese in conto capitale, per 4.740 milioni. In sintesi, le variazioni proposte con il provvedimento in esame denotano una contrazione delle entrate finali pari a 32.091 milioni; la diminuzione delle entrate tributarie riguarda sia le imposte dirette che quelle indirette; appaiono di entità significativa le modifiche riguardanti l'IRE, l'IRES, l'IVA, l'imposta sostitutiva e l'accisa sui prodotti energetici; si riscontrano invece aumenti con riferimento al consumo dei tabacchi e al settore dei giochi. Anche in termini di cassa le previsioni assestate comportano un peggioramento dei saldi. Il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, passa infatti da 79.053 milioni della legge di bilancio

In corrispondenza con il saldo netto da finanziare, peggiora significativamente anche l'avanzo primario, nella misura di 49.031 milioni. Va detto che esiste una correlazione tra tale incremento delle dotazioni di cassa e la misura contenuta all'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, che affronta la problematica della tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disciplina prevista stabilisce, relativamente al pregresso, che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dichiari liquidabili i residui nei limiti delle risorse rese a tal fine disponibili con la legge di assestamento. Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame fissa un limite pari a 90.100 milioni di euro, con un aumento di 67.100 milioni di euro rispetto all'importo determinato nella legge di bilancio che lo indicava in 23.000 milioni. Dalle cifre emerge quindi con evidenza l'effetto negativo della congiuntura in atto sul gettito atteso. Come è infatti noto, l'andamento dell'economia risulta particolarmente rilevante ai fini dell'analisi dell'analisi dell'andamento proprio del gettito delle entrate tributarie. È chiaro che l'analisi della dinamica del gettito che si attende nell'anno in uno siffatto scenario di crisi, relativamente alla distinta e separata individuazione della componente congiunturale della flessione del gettito, rispetto ad altri fattori, quali gli effetti dell'azione amministrativa di lotta all'evasione e all'elusione, non potrà disgiungersi anche dal distinto computo dell'effetto che specifiche misure legislative di politica tributaria avranno nel potenziare gli accertamenti e le riscossioni, ovvero l'eventuale grado di adesione spontanea da parte dei contribuenti. Consentitemi di concludere rilevando come proprio a fronte del calo delle entrate occorra accelerare l'azione di miglioramento della qualità della spesa pubblica. Tale processo richiede la conoscenza dei meccanismi che la regolano e l'individuazione degli innumerevoli fattori che possono comprometterne la realizzazione. Risulta imprescindibile la valutazione di efficienza ed efficacia della spesa pubblica, sia pure con i dovuti limiti per la peculiarità dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica. Anche il settore pubblico dovrà dotarsi, come previsto dalla legge n. 15 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, di una serie di idonei indicatori di *performance*, in modo tale da poter misurare al meglio i risultati effettivamente conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati e delle risorse impiegate allo scopo. Ciò rende altresì necessario valutare l'opportunità di iniziare una seria riflessione sulle modalità di finanziamento di alcune tipologie di servizi al cittadino, soprattutto quelli a domanda individuale, in modo tale da attribuire una maggiore autonomia economica ai cittadini, alle famiglie e alle imprese e, nel contempo, ridurre il peso dello Stato quale soggetto intermediario del sistema. La riduzione del finanziamento dei servizi a domanda individuale da parte dello Stato può consentire ai cittadini di accedervi in maniera autonoma grazie alla maggiore disponibilità finanziaria creatasi per effetto della riduzione dell'intervento pubblico nell'economia. Un'ultima annotazione concerne il ruolo dello strumento della legge di assestamento. La riforma della normativa di contabilità ora all'esame della Camera dei deputati, della quale tutti auspichiamo una sollecita approvazione, rende questo strumento facoltativo e non più obbligatorio, nell'auspicio che una sempre migliore programmazione della finanza pubblica renda la fase di assestamento una necessità sempre più eventuale.

il Governo non sta governando la crisi, ma ne viene governato. Altro che grande ritorno della politica dopo anni di offuscamento e di ridimensionamento del suo ruolo ad opera dell'economia, di cui

ha insistito nel programmare, non prendendo atto che questa era la tendenza, una politica fiscale restrittiva in un clima di profonda recessione. Noi

momento che la manovra è triennale, nel 2010 e negli anni seguenti attraverso riforme incisive dal lato della spesa, da approvare immediatamente nel corso del 2009, in modo da rassicurare i mercati finanziari

meno stupida di quella adottata dall'Unione monetaria europea negli anni precedenti. Il Governo rifiutò questo approccio. Non abbiamo nulla da cambiare della manovra triennale di luglio, ci si disse durante la sessione di bilancio, nemmeno per ciò che riguarda il primo anno e dunque il 2009. In secondo luogo, ci si disse che il debito pubblico è troppo alto per permettersi una manovra espansiva, per quanto responsabile e limitata, e da ultimo ci si disse che non era possibile prevedere riforme strutturali durante la crisi. Fummo facili profeti nel replicare: non volete fare nulla per tentare ora di governare la crisi, lascerete quindi il Paese in balìa della crisi stessa, esposto a pagare un prezzo doppio: subito, quello di una crisi che potrebbe sia pure marginalmente essere resa meno profonda e meno pesante socialmente da un intervento pubblico che aggiungesse una componente discrezionale all'azione degli stabilizzatori automatici; domani, il prezzo ancora più salato di una ripresa che a crisi globale terminata - perché terminerà la crisi globale, come sono terminate quelle che l'hanno preceduta - sarà per noi più debole e stentata, a causa delle mancate riforme strutturali che proprio la crisi rende più urgenti e anche, paradossalmente, più facili politicamente da realizzare, perché rendono meno forti le resistenze conservatrici. In sostanza, dicemmo: non volete cercare di governare la crisi e ne sarete governati; la finanza pubblica peggiorerà, ma non in funzione di un consapevole progetto di sostegno dell'economia, organizzato attorno ad un preciso ordine di priorità economiche e sociali. Sono passati pochi mesi, signor Presidente, e il Governo ha presentato il disegno di legge che stiamo discutendo. E cosa leggiamo nell'assestamento? citare qualche dato. È stato ricordato, tra l'altro, incredibilmente, nella relazione, attribuendo questi dati all'andamento macroeconomico dell'economia, quando è del tutto evidente che, al massimo, è dal lato delle entrate che ci sono effetti sul bilancio indotti dalla crisi, ma dal lato delle spese siamo in presenza di una componente

la legge di bilancio fissa il saldo netto da finanziare in 32,7 miliardi di euro: lo sa, signor Presidente, che adesso, con l'assestamento, il saldo netto da finanziare passa a 69,6 miliardi di euro? che il saldo netto da finanziare, rispetto alla legge di bilancio in vigore, più che raddoppia. Non è mai accaduta una cosa di questo tipo!

L'avanzo primario passa da 48,5 miliardi, come fissato dalla legge di bilancio, a 8,5

Questa, signor Presidente, non è una legge di assestamento: questa è un'altra legge di bilancio! Tutto ciò pone due problemi, uno di forma e uno di sostanza, entrambi serissimi.

può disporre scelte discrezionali di spesa (perché di questo si tratta, dato che il peggioramento dei dati macroeconomici qui non c'entra assolutamente nulla) ed un peggioramento con effetti diretti sul fabbisogno e sull'indebitamento di questa entità,

La risposta è chiara, signor Presidente: assolutamente no, la legge di assestamento non può realizzare un'operazione di questo tipo, se vuole rispettare la legge di contabilità. Non valgono in proposito i precedenti che pure vengono citati del 2008, del 2007 e del 2006; casi questi in cui l'assestamento registrava l'aumento delle entrate rispetto alle previsioni e fissava nell'assestamento degli spazi finanziari che consentivano l'utilizzo in termini di riduzione della pressione fiscale applicando il comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria di tutti quegli anni. quegli anni. Come lei sa bene, purtroppo, e come il relatore ha perfettamente documentato, questo disegno di legge di assestamento non non registra soltanto le minori entrare determinate dall'andamento macroeconomico, ma dispone maggiori spese discrezionali per almeno un punto di prodotto interno lordo ciò che certamente non può essere disposto in base alla legge di contabilità dall'assestamento. Ma perché il Governo ricorre ad una così macroscopica violazione della legge n. 468 del 1978? È chiaro! Premuto da tutti i lati, da emergenze sociali, economiche, territoriali e privo - perché ha rifiutato la proposta che gli abbiamo avanzato un anno fa - di un progetto che gli consenta di ordinarle secondo trasparenti priorità, il Governo cede disordinatamente a queste pressioni e crea uno spazio finanziario, specie dal lato della cassa, che poi cercherà di gestire attraverso la gestione della spesa. E lo fa con l'assestamento e non come avrebbe dovuto con una manovra correttiva del bilancio esplicita perché questo strumento è da sempre politicamente poco impegnativo ed infatti, come vedete, lo stiamo discutendo nella totale disattenzione generale. Il vero problema è che questa è la legge di bilancio e non di assestamento. Ma ecco il secondo problema, signor Presidente, quello di sostanza. Attraverso questa assurda procedura il Governo fa quello che aveva rifiutato di fare soltanto sette mesi fa, cioè una manovra espansiva discrezionale per un punto di prodotto interno lordo, esattamente la dimensione che gli avevamo proposto un anno fa, ma scegliendo la peggiore delle strade possibili dal punto di vista degli interessi del Paese: quella di usare questo punto di prodotto per incrementare la spesa pubblica così com'è, senza alcun ordine di priorità. E noi tutti, signor relatore, signori del Governo, di centro-sinistra e di centro-destra, abbiamo sempre detto che la spesa, così com'è, non alloca le risorse pubbliche in modo efficiente e nemmeno in modo socialmente giusto. Possiamo avere, ed in effetti abbiamo, una diversa visione degli interessi del Paese e della buona allocazione delle risorse, ma gli uni e gli altri sappiamo che una strategia meramente incrementale della spesa, lasciando l'ordine delle priorità attuali, è nemica della buona politica. Questo assestamento è nemico della buona politica. Di qui la proposta che avanziamo: il Governo ritiri il disegno di legge di assestamento, o qui o durante la discussione alla Camera. Questo solo fatto, signor Presidente - attendo di essere confutato dal Governo su questo punto questo punto - migliorerà i dati di finanza pubblica per almeno un punto di prodotto interno lordo. Creerà degli spazi finanziari all'interno dei quali il Governo potrà proporre una discrezionale manovra espansiva di finanza pubblica ancora negli ultimi mesi del 2009, da compensare negli anni successivi. Naturalmente avremo visioni e proposte diverse sui contenuti di questa manovra ma saremo tornati alla politica trasparente, ad un confronto trasparente tra soluzioni diverse e non al ricorso all'inganno, alla violazione delle regole per fare quella manovra surrettiziamente, a seguito dei dettami della crisi stessa, che voi avete negato di fare consapevolmente un anno fa. Infine - e ho terminato, signor Presidente - un'osservazione puntuale che la pregherei di registrare per riferirne anche al Presidente del Senato.

il decreto-legge n. 39 del 2009, all'articolo 14, usa da 2 a 4 miliardi di euro per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, chiediamo al Governo conto dell'avvenuto trasferimento delle risorse in questione dal FAS

(anche qui come si dice dalle mie parti), allora ce ne siamo stati, signor Presidente: abbiamo pensato ad un atteggiamento in buona fede, ad un piccolo ritardo. Ma ora i mesi sono passati ed è arrivato l'assestamento.

Quindi, signor Presidente, c'è una legge che istituisce quel Fondo e lo dota di 9 miliardi di euro, c'è una legge che copre su quel Fondo per 4 miliardi di euro il provvedimento sul terremoto, ma nel bilancio il Fondo non c'è e non c'è nemmeno adesso che è stato presentato l'assestamento, che avrebbe dovuto registrare le variazioni determinate dalle modificazioni legislative intervenute. La mia opinione, signor Presidente (è qualcosa di più di un'opinione, naturalmente), è che il Governo Governo deve - non può - presentare un emendamento all'assestamento per spostare trasparentemente le risorse dal FAS al Fondo strategico e scrivere questo trasferimento in bilancio. Perché il Governo non vuole farlo?

nel Fondo per le aree sottoutilizzate di risorse utilizzabili per lo sviluppo del Sud - lo scopo cui è ordinato il Fondo per le aree sottoutilizzate - non ce ne sono più.

è messo interamente a carico delle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia. Se si trasferiscono i fondi dal FAS al Fondo strategico questa realtà risulta evidente, ammesso che quelle risorse siano sufficienti, ed a mio giudizio non lo sono. Capisco l'imbarazzo del Governo di fronte alla verità dei fatti, una verità così cruda. Se l'imbarazzo è sintomo di consapevolezza merita rispetto, un tentativo di nascondere la verità al popolo italiano in tema di decisioni di bilancio, merita la più assoluta esecrazione e reclama una riparazione. Chiedo formalmente che a questa riparazione si provveda. *(Applausi dai Gruppi PD e

l'assestamento di bilancio per il 2009 evidenzia, come è appena stato ricordato, un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a 36,8 miliardi di euro, attribuibile alla rilevante diminuzione delle entrate per oltre 32 miliardi di euro e ad un aumento delle spese finali di 4,5 miliardi euro. Il calo delle entrate per il 2009 rimane evidente; parliamo di 32 miliardi di euro che verranno a mancare alle casse dello Stato, a fronte della previsione fatta al riguardo alcuni giorni fa dal Presidente del Consiglio, che aveva parlato di un calo delle entrate di oltre 37 miliardi. Tuttavia, si parla sempre di un ingente quantitativo di risorse che, venendo a mancare, comporteranno una riduzione del PIL - e per fortuna il Governo ne ha preso atto - del 5,2 La Relazione unificata sull'economia e la finanza, in contrasto con i dati della Banca d'Italia, ha previsto per il 2009 una riduzione delle entrate tributarie per soli 5 miliardi di euro, con ciò evidenziando la mancanza di una visione reale dell'andamento dell'economia e della finanza pubblica da parte del Governo. Parte di tali minori entrate sono, invece, certamente imputabili ad una forte ripresa dell'evasione e dell'elusione fiscale, come tra l'altro dimostrano i più recenti ed eclatanti risultati conseguiti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate nello svolgimento della propria attività di accertamento e repressione dell'evasione. Il Governo, signor Presidente,

non ha ancora presentato al Parlamento la relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale che, in base all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, doveva essere presentata entro il 30 settembre 2008.

Ma è un recupero arduo perché chi evade ha spesso la certezza dell'impunità e l'ammirazione sociale, perché gli evasori vengono giudicati come tanti furbi da imitare. Infine, la reiterazione dei condoni. Oltre allo scudo fiscale si annuncia il condono tributario per gli ultimi tre anni, tanto che i commercialisti invitano i propri clienti a non pagare le tasse per il 2008. Il Ministro dell'economia si vanta di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma allunga una mano per elemosinare quello che gli evasori ritengono di versare per mettersi in regola con la giustizia fiscale e con quella penale. Esaminando gli aumenti relativi alle spese finali in termini di competenza si tratta di dover sostenere nel 2009 maggiori entrate per 4 miliardi e 457 milioni di euro nell'ambito delle quali spiccano alcune voci, come (l'abbiamo detto più volte in questa Aula): i rimborsi ai Comuni per il minor gettito derivante dall'ICI sui fabbricati rurali che peseranno per 1,5 miliardi di euro, l'adeguamento dei fondi per spese obbligatorie per 300 milioni Per la spesa in conto capitale l'incremento, pari a 6 miliardi e 589 milioni di euro, interessa per 4 miliardi il fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale, 600 milioni le Ferrovie dello Stato e per 150 milioni la contabilità speciale per anticipazione in conto cassa a favore di Alitalia. Altri incrementi riguardano contributi agli investimenti per le amministrazioni pubbliche (400 milioni circa), contributi ad imprese private (300 milioni circa) spese in conto capitale. I numeri di questo disegno di legge registrano il peggioramento - lo voglio ricordare ancora una volta - di 36,548 miliardi del saldo netto da finanziare. Uno dei dati più eloquenti del disegno di legge di assestamento di bilancio è quello che concerne l'integrazione delle autorizzazioni di cassa per circa 18 miliardi, al fine di consentire, come spiega la relazione al disegno di legge, il pagamento di una quota considerevole dei residui passivi iscritti in bilancio e l'accelerazione quindi dello smaltimento dei debiti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Tale dato, infatti, trova riscontro con quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, il cosiddetto decreto Il Governo, quindi, ha inteso chiarire nella relazione che le risorse che dovranno finanziare il pagamento accelerato dei debiti delle amministrazioni verso i fornitori (ovvero,

poiché nell'assestamento ne sono indicati solo 18, mancherebbero all'appello 5 miliardi di euro. È comunque chiaro che nella misura in cui le amministrazioni pagheranno, di altrettanto peggiorerà il fabbisogno ed aumenterà il debito.

Che siano 18 o che siano 23 i miliardi da pagare entro fine anno, di certo c'è solo il fatto che, per la prima volta, vi è la necessità di approvare la legge di assestamento di bilancio prima della pausa estiva. A consuntivo poi si vedrà l'ammontare dei pagamenti effettuati. Per la prima volta, quindi, l'assestamento compie un'operazione di politica economica, aumentando il deficit di cassa. legge di assestamento, che è come il bilancio una legge formale, dovrebbe effettuare in un certo senso manutenzioni del bilancio in corso d'esercizio; di solito non opera variazioni non dipendenti dal ciclo economico. Oggi, invece, ci troviamo di fronte alla seguente situazione: esiste un peggioramento delle entrate per 32 miliardi che l'assestamento registra; il saldo netto da finanziare, però, aumenta di 46 miliardi in termini di cassa.

un deterioramento pesante quello dei conti pubblici nel primo trimestre del 2009: il 9,3 per cento di indebitamento in un trimestre rappresenta un primato negativo almeno dal 1999. Quest'anno poi la recessione economica ha colpito duramente: il PIL del primo trimestre 2009 è sceso, in valore assoluto, da 379,3 miliardi a 367,7 miliardi dello stesso periodo del 2008, ovvero di oltre il 3 per cento; le entrate totali calano, le spese raddoppiano. La spesa della pubblica amministrazione cresce, le entrate fiscali rallentano e lo stato di salute della finanza statale peggiora: questa è la reale fotografia dello stato dei conti pubblici, questo è lo scenario. Non basta l'ottimismo del Ministro dell'economia e delle finanze che continua a dire che la situazione è perfettamente gestibile. L'Italia dei Valori non può nascondere la testa sotto la sabbia: dobbiamo dire la verità al Paese! Siamo molto preoccupati per lo stato dell'economia del Paese, che in parte dipende - come abbiamo evidenziato più volte in quest'Aula - dall'avidità dei banchieri e dalla grave crisi economica, ma dipende anche da politiche economiche sbagliate. Noi ci rallegriamo

parla di trasparenza e di legalità, ma poi si presenta il terzo riciclaggio di Stato a favore di evasori, di contrabbandieri, di trafficanti di armi e droga,

vizioso che non è perfettamente gestibile. Avevamo chiesto di dare il nostro contributo, ma purtroppo questo Governo è abituato a fare strame del Parlamento:

dopo che un cittadino marocchino aveva chiesto di essere assunto all'ATM di Milano e aveva visto respingere la sua domanda in base ad una legge del 1931.

Il Governo non ha minimamente risposto e oggi questo avvenimento, che rappresenta un fatto grave ad avviso mio e dei 30 colleghi firmatari, assume una gravità ulteriore perché la magistratura ha disposto ha disposto l'assunzione del cittadino marocchino. Un noto europarlamentare si si è espresso con parole durissime nei confronti del provvedimento del magistrato, definendolo aberrante e sollecitando i magistrati stessi ad andare a fare il loro lavoro in Marocco. aggiunto che gli autobus italiani, gli autobus dell'ATM, devono essere guidati solo da cittadini italiani. prego la sua cortesia se, con tutta l'autorevolezza che deriva dalla sua alta carica, ella vorrà sollecitare il Governo a fornire

tipo di strategia ha questo Governo in tema di integrazione dello straniero. *(Applausi

Presidente, onorevoli colleghi, il presente intervento non è finalizzato a sollecitare un atto di sindacato ispettivo cui non è stata data risposta, come troppo spesso i senatori di maggioranza e di opposizione debbono fare; si tratta, invece, di segnalare alla Presidenza del Senato la circostanza che interpellanze ed interrogazioni ricevono talvolta risposta, ma con modalità e contenuti tali da far seriamente dubitare del fatto che gli uffici ministeriali preposti leggano e trattino con serietà ed attenzione i quesiti che vengono loro posti dai parlamentari.

che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile scorso, risulta in molti punti imprecisa, se non fuorviante. Non solo gran parte della risposta si limita a riprendere, parafrasandolo, quanto scritto nella premessa ma al primo punto della risposta l'interrogante viene informato dal Governo dell'avvenuto inserimento nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dell'articolo 1-*bis*, volto a cancellare l'ultima proroga delle norme antisismiche sulle costruzioni voluta dal Governo Berlusconi. Tale ottima decisione, solo parzialmente affinata dal relatore in Assemblea, in realtà scaturisce dall'emendamento 1.0.1 del Gruppo dell'Italia dei Valori, a prima firma del senatore Russo e da me cofirmato, approvato dalla Commissione ambiente del Senato. Siamo pertanto grati al Governo di avercela gentilmente ricordata, ma possiamo assicurare di averla avuta da sempre ben chiara. La cosa strana è che nel prosieguo della risposta venga ampiamente citato come modello di prevenzione antisismica cui il Governo intende ispirarsi, in risposta ai quesiti sollevati, il contenuto dell'articolo 11 del decreto-legge sull'Abruzzo: contenuto assai dettagliato e stringente, che oggi però non esiste più in quanto il medesimo Governo lo ha completamente riformulato e snaturato in sede di conversione n. 77). In sostanza, da una parte si dà conto di una modifica apportata dal Parlamento, dall'altra non si dà conto di una contemporanea modifica che peraltro ha praticamente svuotato il severo piano di adeguamento antisismico voluto dal sottosegretario Bertolaso, dando ad intendere che esso sia rimasto invariato. Tuttavia - e mi accingo a concludere - tale modifica è avvenuta in Senato, e noi la conosciamo. Non è certo il caso più grave, dal momento che almeno una risposta c'è stata, ma ho voluto citarlo, signor Presidente, solo in quanto esempio di tante altre risposte che lasciano l'interrogante insoddisfatto in quanto non affrontano puntualmente le domande poste nell'atto di sindacato. Mi rivolgo quindi alla Presidenza perché, tutelando la dignità del Senato, sensibilizzi il Governo non solo a rispondere alle interrogazioni, cosa certo apprezzabile, ma possibilmente a farlo

che, al di là dei Governi e delle maggioranze, esista per il Parlamento italiano un problema che riguarda l'efficacia degli strumenti ispettivi e che esista una cultura del controllo, che è fondamentale in tutti i Parlamenti, che nel nostro Paese, per motivi anche storici, è trascurata e sentita come

Purtroppo, al di là dei momenti di commemorazione, credo che spetti a quest'Assemblea cercare di impedire che tali fatti ormai troppo frequenti si ripetano. Io e altri colleghi del mio Gruppo siamo stati sollecitati in questo senso, prima ancora di questo episodio, dai comitati dei parenti delle vittime delle stragi del 2003 (non so se lei ricorda la strage di Milano di via Carcano e quella di Aci Castello) proprio per intervenire su una legislazione ormai vecchia e incongruente, affinché si limiti la concessione del porto d'armi, rendano più seri e rigorosi i controlli nel periodo della detenzione del porto d'armi stesso (sia che si riferisca a quello per difesa personale, in alcuni casi, che a quello legato alla pratica della caccia) e, soprattutto, si introducano elementi di

la Presidenza farà presente alla Commissione a cui è stata assegnato l'esigenza e l'importanza di una sua calendarizzazione. **Sull'assenza

«Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari (...). Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due». Ebbene, signor Presidente, è un anno che questo Regolamento o non lo abbiamo capito o non è stato

il presidente Schifani in merito all'assenza di un partito che - lo ripeto - è il secondo partito di quest'Aula e del centrosinistra e il quarto partito in Italia? Che cosa ha riferito il presidente Schifani al Presidente della Repubblica? Se ha riferito che è stato composto un Consiglio di Presidenza,

Presidente «sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato». Noi, da un anno a questa parte, non possiamo intervenire sul buon andamento dell'Amministrazione del Senato. Dirò di più le attribuzioni dei Segretari: essi «sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete». Signor Presidente, anche questo ci fa indignare, perché noi non partecipiamo né alle sedute pubbliche né a quelle segrete,

12, il Consiglio di Presidenza «nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi

Presidente, anzitutto la ringrazio della sua cortesia, nonostante l'ora. Vorrei restasse agli atti ed informare l'Assemblea di quanto accaduto lo scorso 17 luglio nel Lecchese, che è stata interessata da due gravi perturbazioni che hanno causato smottamenti e uscite dall'alveo di torrenti e del fiume Rio Torto, provocando la morte di una persona e numerosi sfollati. In particolare, i Comuni di Lecco, Civate e Valmadrera hanno subito danni ingenti e numerose aziende hanno dovuto cessare l'attività, che non è ancora ripresa come lei può capire - in una situazione di crisi già esistente. Già nella giornata di sabato 18 luglio il Presidente della Regione Lombardia, onorevole Formigoni, il Presidente della Provincia ed i tre sindaci dei Comuni interessati hanno chiesto unanimemente al Governo il riconoscimento Ieri oltre 30 senatori del mio Gruppo hanno presentato una interpellanza urgente al Presidente del Consiglio dei ministri. In questo momento il riconoscimento della calamità naturale è urgentemente

un colpo che ha aggravato la pesantezza della situazione economica. Per quanto riguarda la sua richiesta, la risposta spetta alla valutazione dei provvedimenti che saranno portati all'attenzione del Senato,